Colleghi, comunico che è stata trasmessa copia del seguente decreto: «Il Presidente della Repubblica, VISTO l'articolo 86, primo comma, della Costituzione; CONSIDERATA la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprenderà all'estero a decorrere dal 23 ottobre 2010, recandosi nella Repubblica Popolare Cinese in visita di Stato; DECRETA: Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 23 ottobre 2010 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascerà l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

In conseguenza della situazione costituzionale così determinatasi, il Presidente del Senato mi ha incaricato di esercitare per tutto il periodo della supplenza le funzioni di Presidente del Senato in base alla designazione effettuata in data 23 giugno 2008, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del Regolamento. Presidente, il 22 ottobre è pervenuta al Senato una nota del Capo dello Stato

Senatore Belisario, non si può chiedere alla Presidenza di dare lettura di una lettera del Presidente della Repubblica indirizzata non alle Camere, ma al Presidente della 1a Commissione permanente. Mi risulta che il presidente Vizzini abbia letto la lettera oggi pomeriggio ai componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione affari costituzionali e che in tale sede i rappresentanti dei Gruppi si siano impegnati a non discutere della lettera in quanto tale, ma solo delle questioni inerenti l'*iter* del disegno di legge costituzionale. Così è avvenuto anche nella successiva riunione della Commissione plenaria. L'orientamento emerso in Commissione mi sembra corrispondere pienamente a criteri di correttezza e rispetto dovuti al Presidente della Repubblica. intervengo innanzi tutto per ringraziarla per la valutazione che ha testé espresso del comportamento tenuto in Commissione affari costituzionali nei confronti della lettera inviataci dal Presidente della Repubblica. Voglio soltanto precisare che a seguito della lettura della lettera non solo non si è aperto alcun dibattito sulla lettera stessa, per i motivi che lei stessa ha voluto citare, ci sono stati degli interventi sull'ordine dei lavori alla fine dei quali si è convenuto di riaprire i termini per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in oggetto sino alle ore 16 di giovedì.

Questo è quanto è avvenuto in Commissione, né altro poteva avvenire su una lettera come quella inviata dal Presidente della Repubblica.

con la quale sono stati calendarizzati per domani pomeriggio la discussione e il voto di proposte di risoluzione o altri documenti relativi alla riforma riforma della *governance* economica e di bilancio dell'Unione europea - il cui esame è oggi iniziato presso la 5a Commissione - e di una mozione sulla politica economica presentata dal senatore Rutelli

lo svolgimento di un'unica discussione, dopodiché saranno presentate le risoluzioni, come disposto dalla Conferenza dei Capigruppo, relativamente a questa importantissima materia che è la riforma sul coordinamento europeo delle politiche di bilancio, allora va bene. Se invece si intendesse ugualmente dare corso a due votazioni distinte, due votazioni distinte, dovrebbe essere allora disposta una separazione della trattazione dei due argomenti, perché esiste sì una qualche connessione tra le due materie, ma molto indiretta. Un conto infatti è la discussione e l'esame dei documenti dell'Unione europea

chiarimento su questo punto per poter meglio ordinare i nostri lavori. Ove la Presidenza dovesse ritenere di separare queste discussioni, come io auspicherei per ragioni di ordine e di chiarezza, sarebbe altresì auspicabile, in relazione alla necessità di avere qualche ora in più di discussione su una materia così importante come quella europea, differire l'esame e il voto delle risoluzioni a giovedì mattina, cosa che peraltro non comporterebbe alcuno stravolgimento del calendario, perché fino a giovedì mattina è possibile concludere l'esame di questi argomenti. La pregherei pertanto ordinare la nostra discussione secondo quanto ho rappresentato. la Conferenza dei Capigruppo, nella riunione svoltasi in pari data, ha stabilito, con decisione unanime, su proposta del rappresentante del Gruppo del Partito Democratico, di inserire nel calendario dei lavori un dibattito con riferimento a schemi di regolamenti comunitari su procedure di sorveglianza e coordinamento delle politiche economiche europee, all'esame della 5a Commissione permanente. Nell'ambito di tale dibattito, che costituisce l'oggetto principale della discussione, è stato poi chiesto, su proposta di altri Gruppi, di assorbire anche la mozione Rutelli ed altri in materia di politica economica. Questo è pertanto quello che prevede il calendario adottato all'unanimità dalla Conferenza dei Capigruppo.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, oggi nell'Aula del Senato ci si confronta su una questione di grande rilievo per il futuro dell'agricoltura, che riguarda non solo i 13.600.000 occupati nel settore in Europa, ma ben 500 milioni di consumatori interessati al mantenimento delle capacità produttive del sistema alimentare europeo e alla qualità dei prodotti, su cui sempre di più chiedono di conoscere ed esprimersi, decidere.

Per questo il Gruppo PD ha fortemente voluto un confronto in Aula sul futuro della riforma della politica agricola comune, cioè la PAC oltre il 2013. La Commissione europea presenterà la comunicazione con le linee strategiche entro il mese di novembre. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in merito. Il commissario Dacian Ciolos ha promosso una grande consultazione aperta al contributo di tutti i cittadini europei conclusasi il luglio scorso. Il Parlamento italiano non può essere assente in questo dibattito; dunque siamo contenti che sia stata accolta la nostra sollecitazione. Il confronto sul futuro della PAC per il nostro Paese è questione di grande rilievo: stiamo parlando di risorse che oggi per l'Italia ammontano a 6 miliardi di euro e che, dobbiamo saperlo, rischiano di diminuire drasticamente se si andrà verso scelte che prevedono livellamenti burocratici della distribuzione delle risorse, risorse, con ripercussioni pesanti sulla tenuta sociale dei territori, della loro identità. Parliamo - in estensione - del 50 per cento di questo Paese e di quasi la totalità dei territori del Sud Italia; parliamo di sicurezza alimentare e di salute, fino a nuovi sistemi di produzione energetica: questa è la nuova dimensione e la grande valenza dell'agricoltura nel mondo contemporaneo. Questione non più settoriale, ma centrale e come tale incrocio di grandi contraddizioni e criticità opposte che procedono in parallelo: emergenza alimentare per oltre un miliardo di persone e nello, stesso tempo, spreco di alimenti fino al 30 per cento nel sistema alimentare; emergenza obesità in crescita nel mondo occidentale; bisogno di maggiore produzione di cibo, da un lato, superfici agricole che diminuiscono, perché utilizzate diversamente e sottratte alla produzione di cibo, Un mercato che domanda più cibo di migliore qualità e, nello stesso tempo, vede il reddito dei produttori in calo, in continua diminuzione: meno 12,2 per cento la media europea (meno 25 per cento nel nostro Paese). L'agricoltura italiana, del resto, è esempio emblematico di queste contraddizioni: ha forte potenzialità, è patria delle diversità produttive agricole pregiate, ha una vocazione riconosciuta nel mondo e, insieme, forti limiti e problemi propri di un sistema agroalimentare che abbiamo radiografato più volte (eccessiva frammentazione, carenza organizzativa, irrazionalità logistiche, inefficienze nelle filiere alimentari, che portano ad una squilibrata distribuzione del valore, ad una burocrazia eccessiva vuota di significato e carica di costi). Ma una grande parte dei problemi deriva anche da fattori esterni non governabili dai produttori, come le emergenze climatiche in crescita o le distorsioni mondiali dei prezzi, che portano a volatilità così forti in tempi tanto brevi da non poter essere affrontate dentro le logiche delle normali dinamiche di mercato. A monte di tutto questo, l'Italia agricola soffre oggi di un problema ancor più grave: la scarsa considerazione sociale, oltre alle difficoltà economiche di chi produce cibo. Una marginalità della professione che allontana i giovani e non intercetta le loro aspirazioni: basti pensare che solo il 7 per cento degli imprenditori al di sotto dei 40 anni è impegnato nel settore ed un processo di modernizzazione non può certo avvenire senza un ricambio ed una forte qualificazione del capitale umano, senza nuove competenze, nuovi saperi, ma anche nuove modalità di integrazione. un inserimento utile e prezioso dei lavoratori stranieri nel settore, un intervento organico e non legato alle improvvisazioni, allo sfruttamento ed all'illegalità. Per questo motivo nei meccanismi incentivanti il parametro «lavoro regolare» la sua tracciabilità sarà questione decisiva. una nuova capacità di fare impresa. Di questo ha assolutamente bisogno il sistema agricolo europeo, il sistema italiano in particolare, perché sia in grado di governare e non subire la profonda trasformazione che è avvenuta con l'apertura dei mercati a livello globale in cui, al tempo stesso, entrano nuovi potenti concorrenti e, per la prima volta, entrano grandi masse di nuovi consumatori o vecchi consumatori con nuovi bisogni. Per questo, affrontare il tema della PAC e del suo futuro significa partire dal riconoscere la grande trasformazione in atto, riconoscere che l'attuale sistema della PAC è ormai inadeguato, perché non risponde più alle esigenze di un settore che aspira ad essere motore trainante dello sviluppo europeo. Occorre introdurre più dinamicità, più protagonismo ed autonomia dei produttori, nuovi fattori di competitività. Dobbiamo avere il coraggio di dire che l'attuale PAC non è abbastanza proiettata su questi obiettivi, che è una politica troppo rivolta al passato. Occorre passare da una politica di sostegno e di premialità alle posizioni di rendita (ovvero la proprietà della terra, la titolarità dell'azienda, i diritti acquisiti e mantenuti in modo statico) alla concessione ed incentivi per precisi comportamenti. Come ben riportato dal rapporto INEA, patrocinato dal Ministero delle politiche agricole, occorre introdurre nuovi parametri di valutazione che prevedano, oltre alla qualità ambientale, valore e qualità delle produzioni, capacità di impresa, più efficienza, più innovazioni di prodotto e di processo, capacità di fare sistema dentro la filiera, capacità di creare occupazione qualificata e regolare: questo va premiato ed incentivato. Se si vuole davvero uscire da logiche di assistenza, da una marginalità senza ritorno, la politica per i sistemi agricoli ed alimentari deve promuovere lo sviluppo di imprese agricole sempre più capaci di rapportarsi sul mercato. Per questo una buona politica deve far funzionare i mercati, non sostituendosi ad essi ma cercando di regolarli prevedendo parametri chiari, norme condivise, sistemi di controllo efficaci e sanzioni tempestive che contrastino contraffazioni ed ogni forma di illegalità.

valorizzare le produzioni di qualità, senza penalizzare altri Paesi, senza farsi tentare da politiche neo protezioniste. Ma c'è un beneficio pubblico che il mercato non riconosce; quella produzione di servizi pubblici che riguarda il mantenimento della qualità del suolo e la salvaguardia delle specie animali e vegetali, quell'agricoltura (soprattutto quella a bassa intensità) che concorre alla conservazione del patrimonio paesaggio (dai vigneti, al bosco, agli ulivi, alle coltivazioni a terrazza, ai pascoli d'alta quota). Qualcuno le ha definite le agricolture eroiche, di cui tutti usufruiscono, di cui tutti i cittadini possono beneficiare. Riconoscere valore pubblico al bene pubblico creato dall'agricoltura è un dovere, è giusto, e se andiamo a ben vedere, è un risparmio anche per lo Stato che dovrebbe addossarsi costose manutenzioni territoriali. Se fatto su ambiti definiti, con criteri misurabili non si traduce in assistenza, in attese passive, ma in incentivi al mantenimento dei suoli e delle acque e della specificità dei singoli territori: elementi preziosi per avviare nuove sfide competitive dei territori rurali, per rispondere a nuove domande legate al bisogno di natura, di salute, di autenticità di produzione e di colture. Significa creare migliori condizioni per il futuro e la vitalità dei territori, nuovamente capaci di attrarre generazioni più giovani, più donne imprenditrici (potenziale prezioso ma inespresso), per fare inclusione sociale. Una scommessa dell'agricoltura molto ambiziosa, un modello tutto europeo del tutto inedito che potrebbe fare incontrare redditività e beneficio pubblico: fare impresa nel far bene all'ambiente; fare impresa nel far bene alla salute e nel considerare la dignità e il valore del lavoro. Per tutto questo, nella mozione che presentiamo chiediamo un impegno al Governo perché si faccia promotore di un confronto ampio sulla riforma della PAC con le rappresentanze economiche, sindacali e con le istituzioni, perché il nostro Paese possa presentarsi con una proposta forte nata da una condivisione forte. Chiediamo che si attivi e ricerchi alleanze con i Paesi che rivendicano un *budget* adeguato nel bilancio europeo, indispensabile alle nuove responsabilità che il settore agricolo deve assumere. Chiediamo al nostro Governo che si faccia interprete della visione innovativa di una moderna competitività che punti al rafforzamento della capacità d'impresa, che abbia come motore trainante la conoscenza e l'innovazione e come valori di riferimento irrinunciabili che punti allo sviluppo di reti d'impresa e di azioni di sistema più che di azioni individuali perdenti. Chiediamo che venga dato rilievo e nuove responsabilità alle organizzazioni dei produttori e che si definiscano chiaramente indirizzi, priorità e nuovi obiettivi dello sviluppo rurale. Per quanto riguarda i pagamenti diretti, puntando al mantenimento del *budget* storico del nostro Paese, è indispensabile, per una riconversione vera del nostro sistema, che si ridefiniscano parte dei criteri di assegnazione; che una componente dei pagamenti contempli le differenziazioni territoriali preveda gli svantaggi naturali e ambientali; che preveda il criterio produttivo, tenendo conto delle ricadute occupazionali di intensità e di qualità, e il criterio organizzativo, sia nelle aziende di grosse dimensioni che di dimensioni minime. Queste sono anche le richieste che vengono dalle Regioni, in modo unitario. Nelle misure di mercato, dunque, il presupposto per una prospettiva reale sta nel miglioramento del funzionamento della catena alimentare, nella regolazione dei mercati, nel rafforzamento delle organizzazioni interprofessionali e nell'incentivazione di un'agricoltura contrattualizzata. Ma è assolutamente indispensabile un nuovo sistema di gestione del rischio e nuovi strumenti per affrontare sia la conseguenza delle calamità naturali, sia la creazione di un'opportuna rete di sicurezza contro la volatilità dei prezzi, strumenti in grado di dare risposte rapide ed efficaci alle crisi che sorgono nel settore, quelle imprevedibili e non programmabili. Signora Presidente, questi sono i punti fondamentali riportati nella mozione: diverse considerazioni che, pur con modalità e linguaggi diversi, linguaggi diversi, abbiamo ritrovato nelle altre mozioni depositate. Per questo mi auguro che proprio da quest'Aula oggi possa partire una posizione comune, pur nelle diverse espressioni. Sarebbe un segnale importante per il Governo che si presenta al tavolo europeo e un segnale di speranza e fiducia per gli agricoltori e i consumatori italiani. Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, la politica agricola comune costituisce ancora una delle più importanti politiche dell'intero quadro istituzionale europeo e i suoi obiettivi principali, stabiliti nel Trattato di Roma, sono rimasti pressoché immutati negli anni. Quello che invece si è modificato ed è in continua evoluzione è l'approccio e gli interventi che via via sono stati messi in campo. La politica agricola comune può in un certo senso rappresentare le specchio dei problemi, delle trasformazioni e degli sviluppi di mezzo secolo del nostro continente. Guardando alle sue origini, cinquant'anni fa, appare evidente come la priorità era quello di produrre cibo sufficiente per un'Europa che usciva da un decennio di carestie dovute alla guerra: mangiare ogni giorno era l'urgenza di una politica di ricostruzione e l'agricoltura era quel settore da rilanciare, sostenere e proteggere. Non a caso la PAC è diventata la più importante e la più complessa delle politiche dell'Unione, assorbendo per decenni i due terzi del bilancio comunitario: un impegno finanziario gravoso, utilizzato per creare un mercato unificato, sostenere la presenza dei prodotti europei e proteggerli dalle importazioni e offrire sussidi agli agricoltori tali da incentivare le produzioni. Un impegno che ha prodotto risultati importanti, che ha permesso di mantenere in vita l'agricoltura comunitaria, ma che per contro ha dato il via, sotto gli stimoli degli incentivi, ad una sovrapproduzione incontrollata di alcune produzioni. Per ovviare a ciò, dopo sei anni dalla sua entrata in vigore, nel 1968, si perfeziona il primo tentativo di risolvere i problemi della PAC, che da allora è passata periodicamente attraverso alcune grandi riforme. Penso al Libro verde del 1985, immaginato nell'ottica di ristabilire un equilibrio fra domanda ed offerta, alla riforma MacSharry del 1992, con le misure per la diminuzione dei prezzi agricoli e la protezione dell'ambiente, o ad Agenda 2000, la riforma forse più radicale, che ha preso in considerazione le problematiche economiche, ambientali e rurali nel loro complesso. Con Agenda 2000 infatti all'agricoltura viene riconosciuto, oltre alla funzione produttiva, il ruolo nella conservazione del paesaggio, nella protezione dell'ambiente, nella qualità e sicurezza dei prodotti alimentari e nel benessere degli animali. Viene introdotto il concetto di multifunzionalità e gettate le basi per lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e concorrenziale. Da queste basi ha preso spunto poi la riforma Fischler, quella approvata nel 2003, con la quale viene introdotto il meccanismo del disaccoppiamento degli aiuti, cioè un pagamento unico per un sostegno che il produttore riceve indipendentemente dalla produzione, la modulazione ossia una riduzione lineare degli aiuti della PAC nel corso degli anni, lo spostamento di fondi sul secondo pilastro della PAC, lo sviluppo rurale e la condizionabilità cioè il rispetto delle regole agroambientali (principio "inquinatore-pagatore"). Un percorso che è proseguito negli anni e che, anche nel corso della "valutazione dello stato di salute" della PAC, ha visto un ulteriore ammodernamento della politica agricola comune con importanti risultati anche per il nostro Paese soprattutto nel settore lattiero-caseario. Tutto questo *excursus* per dimostrare la capacità della PAC di sapersi modificare con il tempo, di adeguarsi alle nuove esigenze, ai nuovi contesti, ad un mercato globalizzato e in rapido mutamento. Oggi, come sappiamo, si è già ampiamente avviato il dibattito che porterà al futuro della PAC dopo il 2013. Un futuro che dovrà più che mai tenere conto dei cambiamenti degli scenari economici, che dovrà più che mai tenere conto delle nuove sfide che attendono le imprese agricole europee. L'allargamento dell'Unione, l'aumento della popolazione agricola, delle superfici coltivabili, di quelle rurali, il nuovo potenziale di produzione agricola degli Stati membri impongono scelte efficaci, interventi in grado di contribuire e migliorare la competitività, l'innovazione, la partecipazione alla filiera, garantire redditi soddisfacenti agli agricoltori europei, senza trascurare gli obiettivi legati alla qualità delle produzioni, al rispetto dell'ambiente, alla biodiversità, alle risorse idriche, alle fonti energetiche. Il dibattito europeo sulla riforma ha già fatto emergere la considerazione unanime secondo cui la PAC deve rimanere una politica comune forte, strutturata sui suoi due storici pilastri e improntata a valorizzare il ruolo degli agricoltori, ad avvicinare la produzione agricola ai consumatori e al mercato per rispondere alla crescente domanda di informazione e di trasparenza, e a rafforzare il potere delle imprese agricole nell'ambito delle filiere. Colleghi, tutti sappiamo che l'agricoltura è un malato grave, non solo in Italia, non solo in Europa, ma in tutto il mondo. Una situazione che ha spinto in questi anni i più grandi Governi mondiali a sostenere attivamente e con forza il proprio sistema agricolo. E in Italia, il Paese delle eccellenze agroalimentari, della qualità e della tipicità delle produzioni, l'agricoltura da anni è in crisi profonda, una crisi diffusa che alle difficoltà congiunturali affianca quelle strutturali. Le cifre, i dati, ma soprattutto il dramma sociale del mondo agricolo lasciano poco spazio ad ulteriori commenti. Un dramma vero, un dramma che vede molte famiglie che vivono di agricoltura assestarsi al di sotto della soglia della povertà, non potendo far fronte ai minimi bisogni familiari né, tanto meno, al pagamento dei debiti bancari, dei contributi, né alle spese vive per continuare a lavorare la terra o allevare bestiame. Una crisi silenziosa che spesso passa in secondo piano rispetto a quella di altri comparti produttivi, una crisi che stenta a raggiungere il cuore del sistema e che si impossessa delle pagine dei giornali o delle agende politiche solo quando si riempiono le piazze, si occupano i luoghi istituzionali o peggio ancora solo quando scoppiano gli scandali legati ai suoi prodotti: penso alla mucca pazza, ai vini e oli adulterati, alle coltivazioni OGM o ai sequestri di falsi *made in Italy*. Una situazione inaccettabile per un Paese come l'Italia, che vanta il primato della salubrità e della sicurezza alimentare delle produzioni, una situazione che logora alla base la serenità delle famiglie che con il loro lavoro fanno dell'agricoltura una irrinunciabile colonna portante dell'economia italiana. Una situazione in alcuni casi esplosiva come quella del settore ovi-caprino, come quella di questi giorni in Sardegna dove i presidi dei pastori, le mobilitazioni dei lavoratori delle campagne palesano a tutti noi la drammaticità e il malessere di chi oggi continua a fare quel mestiere che si tramanda da padre in figlio, quel mestiere che non ti fa conoscere né feste né domeniche, ma soprattutto che fa parte della storia, della cultura e dell'economia del nostro Paese. Colleghi, con l'approvazione di questa mozione, vogliamo rafforzare il sostegno e la condivisione con il Governo e con il ministro Galan degli interventi necessari a rafforzare e rilanciare il ruolo dell'agricoltura italiana nel panorama internazionale. Appare infatti più che mai doveroso che il Governo continui nella partecipazione attiva della elaborazione della riforma della politica agricola comune, considerandola un fattore strategico di competitività per tutto il Paese, per il superamento dell'attuale fase di stagnazione economica e di crisi occupazionale. È opportuno, e lo affermo conscio che è già nell'agire del Governo, profondere il massimo sforzo affinché sia mantenuto l'attuale livello di finanziamento della politica agricola comune nell'ambito del bilancio dell'Unione europea, anche in considerazione dell'ampliamento ai nuovi Paesi. Così come occorre adoperarsi per salvaguardare la redditività ed il mantenimento delle produzioni mediterranee, la qualità, l'origine e la tracciabilità delle filiere agricole. Al fine di tutelare e promuovere l'agricoltura italiana andranno altresì previste, all'interno della revisione della PAC, misure specifiche per favorire l'accesso diretto degli agricoltori al mercato, sia attraverso la diffusione dei mercati locali di vendita diretta, sia attraverso il sostegno all'aggregazione delle imprese agricole per consentire l'accesso diretto a mercati più vasti. Bisognerà operare per migliorare la trasparenza del mercato, consolidare una politica della qualità e dell'informazione dei consumatori attraverso la completezza dell'etichettatura dei prodotti e garantire che a livello europeo le importazioni rispettino le norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare e tracciabilità degli alimenti. Il Governo sarà sicuramente in prima linea nel processo di riforma per il dopo 2013, un impegno affinché fra gli strumenti basilari e indispensabili per l'agricoltura italiana vi sia il il mantenimento dell'articolazione della PAC nei due pilastri, vi sia la conferma del pagamento unico aziendale (PUA) in forma disaccoppiata, non più come compensazione, ma come strumento per remunerare i beni e servizi prodotti dagli agricoltori, vi sia una componente innovativa del PUA direttamente erogata agli agricoltori e condizionata al loro protagonismo nelle filiere agricole. Vi siano anche quegli aspetti oggetto dell'integrazione e della modifica al testo della mozione che ho sottoposto all'Aula. concludendo, la situazione di profonda crisi del settore primario implica doverosi interventi: occorre rimettere l'agricoltura al centro delle scelte economiche e della politica, ad ogni livello, dalle azioni che attua ogni singolo Comune, ogni singola Provincia, ogni Regione, alla visione strategica che devono avere il Paese e la Comunità europea. Non dimentichiamoci che l'agricoltura è alla base della nostra civiltà. Non dimentichiamoci che l'agricoltura è alla base del benessere economico e dello sviluppo di ogni Paese.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, questa mozione rappresenta un investimento per il sistema agroalimentare italiano. Essa ha la finalità di sensibilizzare l'impegno del Governo alla tutela della peculiarità dei nostri prodotti,

È nostro dovere, quindi, quello di operare per promuovere la qualità delle nostre produzioni, tutelandole dai tentativi di imitazione e dalla concorrenza sleale, figli di una incontrollata globalizzazione. Il pericolo maggiore è stato, fino ad oggi, quello orientale della Cina. Da qualche anno a questa parte, però, la minaccia proviene anche da Paesi comunitari, soprattutto dall'Europa dell'Est: è di questi giorni la notizia del Parmigiano Reggiano contraffatto prodotto in Romania e di tanti altri esempi negativi di concorrenza sleale che finirà solo con l'approvazione del provvedimento sul *made in Italy* voluto dal nostro ex ministro Zaia. Questi beni rischiano di essere importati in Italia e, conseguentemente, finire sulle tavole dei nostri cittadini: il tutto a loro completa insaputa, in quanto sulle etichette degli alimenti non è obbligatorio indicare il Paese di provenienza della materia prima. Tutto questo a causa di ritardi normativi a livello europeo che continuano a consentire importazioni selvagge (quella cinese è aumentata del 77 per cento) a danno dei consumatori e dei prodotti nazionali. Oggi si possono trovare in commercio prodotti dalla dubbia provenienza e, sempre più spesso, queste derrate alimentari sono reperibili tutto l'anno, indipendentemente dalla loro stagionalità, grazie a trattamenti a cui vengono sottoposti gli alimenti. importante sottolineare come, perché ciò avvenga, essi siano contaminati dai sempre più utilizzati OGM, che rendono le pietanze, forse, esteticamente più belle, ma impoverite dal punto di vista nutrizionale, ricadendo negativamente sulla tradizione italiana della dieta mediterranea, esempio di corretta e sana alimentazione; dieta riconosciuta a livello mondiale come patrimonio immateriale dell'umanità. Come si legge nella mozione che abbiamo presentato, tra gli obiettivi futuri della PAC vi è la sicurezza alimentare, la sostenibilità ambientale e il legame con il territorio. sostenibilità ambientale, che promuoviamo attraverso la valorizzazione dei prodotti biologici e la netta e determinata contrapposizione agli OGM. La sicurezza alimentare, fortemente voluta, nel rispetto della tutela dei consumatori, attraverso il provvedimento il provvedimento sul *made in Italy*. Il legame con il territorio, attraverso la valorizzazione dei 4.396 prodotti tipici delle nostre Regioni. Con orgoglio, la Lega Nord continua a a portare avanti questi suoi cavalli di battaglia, avendo sempre lavorato nel nostro Paese, come in Europa, per la salvaguardia e la promozione della specificità della produzione *made in Italy*.

necessario ed urgente il dibattito odierno sul futuro della PAC, che avviene su sollecitazione del Parlamento. Urgente, perché è noto che nella prima quindicina di novembre l'Italia dovrà intervenire con sue proposte e la PAC rappresenta certamente un interesse notevole per l'Italia, nonostante l'agricoltura europea stia soffrendo e l'agricoltura italiana non sia in buona salute. italiana non sia in buona salute. La politica agricola comune, nata negli anni '50, considerato il contesto conseguente agli eventi bellici, non poteva che essere rivolta essenzialmente al perseguimento dell'autosufficienza nella produzione alimentare. nel Trattato di Roma ci si preoccupò di conciliare le esigenze di due soggetti: gli agricoltori (per garantire loro una remunerazione equa, migliorando il loro reddito individuale, anche attraverso interventi per lo sviluppo del progresso tecnico, l'incremento della produttività, l'impiego migliore della manodopera) e i consumatori, ai quali bisognava garantire sicurezza di approvvigionamenti e, soprattutto, prezzi ragionevoli. L'Europa doveva affrontare subito il fenomeno dell'urbanesimo, legato all'industrializzazione dei territori, con i costi sociali che comportava e la conseguente scelta dell'Europa di una politica costosa per prevenire o comunque frenare l'urbanizzazione delle popolazioni rurali. In rapporto a questo fenomeno, la PAC si assunse l'onere e l'impegno di governare i cambiamenti determinati dal progresso tecnologico, riuscendo a garantire sicurezza alimentare e prezzi elevati agli agricoltori europei, attraverso un tempestivo intervento comunitario, sia sui prezzi, sia attraverso una serie di dazi a compensazione della differenza fra prezzi agricoli europei e prezzi dei Paesi extraeuropei, per evitare flussi eccessivi di importazione. In questo contesto, è evidente l'impegno finanziario comunitario dovesse essere all'epoca molto rilevante, oltre l'80 per cento, ben lontano naturalmente da quello attuale, che deriva dalle numerose riforme della PAC attuate in quattro decenni. Basterebbe ricordare alcune delle tappe, a cominciare dal piano Mansholt del 1968, con la previsione di ridurre la popolazione attiva in agricoltura e l'incoraggiamento alla formazione di unità di produzione agricola più grandi e più efficienti. Gli effetti dello spirito originario della PAC avevano generato in Europa una produzione superiore al consumo: da qui la decisione di concedere sussidi alle esportazioni, per eliminare o almeno ridurre il *surplus* prodotto. Ma con il tempo, gli Stati Uniti e i Paesi in via di sviluppo, lamentando la distorsione della libera concorrenza dei beni agricoli, nell'Uruguay Round (dal 1986 al 1994) chiesero all'Europa di eliminare i sussidi entro il 2000 e, nonostante le vibrate proteste degli agricoltori europei, ottennero che l'Europa cedesse, riducendo i sussidi di un terzo nei sei anni successivi. L'Uruguay Round segna uno snodo fondamentale per la riforma della PAC da parte dell'Europa. Nel 1984, in verità, erano state già introdotte le famigerate quote latte, che tanto hanno penalizzato l'Italia negli anni successivi, in ogni trattativa di politica agricola. Nel 1988, con la riforma Delors, si impose un tetto massimo per le spese agricole e le quote di produzione. Nel 1992, ci fu la riforma MacSharry, con la riduzione dei prezzi garantiti, gli aiuti diretti agli agricoltori, le misure di sostegno per la produzione e l'ambiente. Incominciava a fare capolino l'ambiente, che trovò piena collocazione con Fischler ed Agenda 2000. Anche qui vale la pena di ricordare il contesto politico ed economico in cui si inquadra Agenda 2000: l'avvento dell'euro e il confronto competitivo fra Europa e Paesi in via di sviluppo, situazioni che imponevano all'Europa di non finalizzare la sua politica agricola solo alla finalità tradizionale di produzione di derrate, ma di far diventare l'agricoltura anche guardiana, per così dire, del territorio e fornitrice di servizi per l'ambiente. Si riconosceva, insomma, il ruolo multifunzionale dell'agricoltura, anche a seguito di una giurisprudenza evoluzionista della Corte di giustizia europea, che ha portato all'inserimento nel Trattato di questo ulteriore obiettivo trasversale, tant'è che nel Trattato di Amsterdam del 1997 l'ambiente assurge a principio generale dell'Unione, che deve essere integrato nella definizione ed attuazione delle politiche settoriali comunitarie. Sicché le preoccupazioni legate allo sviluppo sostenibile in agricoltura e all'ambiente trovano adeguato spazio, sia nel primo pilastro (cioè nelle politiche di mercato) sia nel secondo (nelle politiche di sviluppo rurale). È evidente che le finalità della PAC si sono ampliate notevolmente, spaziando dall'ambito economico a quello ambientale e rurale e generando conseguenze sulla PAC stessa e sulle modalità e gli obiettivi di utilizzo del *budget*,

Se è evidente dunque il cambiamento con Agenda 2000, non possiamo non ricordare che nel 2003-2004, con Fischler, si produce un forte cambiamento, con l'introduzione dei pagamenti disaccoppiati, tema oggi all'attenzione dell'*health check* prossimo per gli effetti che ha prodotto. A noi pare che l'attuale PAC sia inefficace ed inefficiente, perché prevede un sostegno ai produttori e non al prodotto, un unico pagamento degli aiuti *pro* azienda indipendente dalla produzione, anche se vincolato alla cosiddetta condizionalità ambientale, un aiuto cioè subordinato al rispetto di una serie di standard di carattere agroambientale, secondo criteri di gestione obbligatori e sulla base del rispetto delle buone condizioni ambientali ed agronomiche. Ma è da considerarsi un fatto positivo che, come effetto dell'aiuto diretto e indipendente dalla produzione, dal 2003 ad oggi siano stati sottratti alla produzione, ad esempio, oltre 300.000 ettari a grano duro? La riflessione sulla validità della riforma risale già a due anni addietro, quando la Commissione presentò la sua proposta di valutazione ponendo diversi problemi: la correzione del regime di pagamento unico; la semplificazione della condizionalità; un sostegno parzialmente accoppiato; lo stabilire un minimo e un massimo di pagamenti, lasciando che i risparmi all'interno di uno Stato potessero essere utilizzati per nuove sfide; l'abolizione del *set aside* per i cereali; il cosiddetto atterraggio morbido per le quote latte; la gestione dei rischi per riorientare la produzione; la lotta al cambiamento climatico, con tutte le implicazioni che comporta in termini di gestione delle risorse idriche e gli interventi sulle colture energetiche. Ma il dato forte di mutamento che emerge dai documenti comunitari è la volontà di rinforzare finanziariamente il secondo pilastro (lo sviluppo rurale), sostenuta dalla Commissione nella sua comunicazione del 18 marzo 2008, e la volontà del Parlamento europeo di conferire aiuti PAC soltanto ai veri agricoltori, ma anche di indicare misure concrete antispeculative, misure di tutela di DOP e IGP, un marchio europeo di qualità, un'etichettatura che contenesse l'origine, delle assicurazioni multirischio. All'epoca, il ministro Zaia si soffermò sulle quote latte (aderendo alla proposta di abolizione nel 2015) e sul mantenimento del premio accoppiato per il tabacco. Forse, sarebbe stato utile appoggiare le richieste dei francesi di mantenere i premi accoppiati nei territori cosiddetti fragili.

primo fra tutti, la redistribuzione fra gli Stati membri, nella prossima riforma, delle risorse destinate agli aiuti diretti disaccoppiati, che giustamente viene indicata come un pericolo, se non è impostata sulla corretta scelta del parametro di riferimento. se si continuasse a pensare al fattore superficie quale parametro unico di ripartizione, si svilirebbe la ricchezza dell'agricoltura comunitaria, che è rappresentata dalla sua realtà multiforme. Noi preferiremmo che l'Italia sostenesse la valutazione di tutti i fattori produttivi, a partire dal capitale e dal lavoro, fino al valore delle produzioni e della professionalità, al mantenimento delle tradizioni, alla sostenibilità sociale ed ambientale. Vorremmo che l'Italia sostenesse gli agricoltori in maniera concreta in presenza di situazioni di crisi di mercato, chiedendo all'Europa una riforma improntata a criteri di sussidiarietà e flessibilità, che consentano di prevenire e quindi di gestire le crisi che si verificano sia in particolari settori, sia in particolari Regioni. Una flessibilità che chiediamo anche per lo sviluppo rurale, attraverso cui si possano gestire unitariamente le risorse assegnate ai diversi programmi regionali. Corretta mi sembra anche l'indicazione da parte di INEA di armonizzare le regole, di agevolare l'integrazione tra fondi strutturali e FEASR. Ma occorre, signor Sottosegretario, che l'Italia, prima di trattare con l'Europa, impari a trattare al suo interno, in forme molto più partecipate delle attuali. Il metodo della consultazione pubblica europea sia adottato anche dall'Italia come buona prassi, così come è giusto che sia. Quanto sarebbero utili, per esempio, anche le consultazioni con le università: quanto sarebbe utile immaginare le università come sostegno organico di consulenza al mondo agricolo per il settore della ricerca. Viene da chiedersi: quante aziende agricole hanno fatto ricorso, ad esempio, al VII programma quadro? Vorremmo poter dire che l'Italia si presenta in Europa con una posizione condivisa,

Purché sia adeguatamente consultato, per tempo, e tenuto in considerazione. Non facciamo che le beghe interne al territorio nazionale debbano pesare negativamente sulle scelte europee. Gli agricoltori italiani meritano molto, molto di più di quanto fino ad ora abbiamo fatto per loro. colleghi, il Gruppo dell'Italia dei Valori vuole approfittare di questo dibattito sulla politica agricola comune, teso a chiedere al Governo impegni precisi in vista della sua riforma, per sollevare problematiche che, a nostro avviso, l'Esecutivo da subito potrebbe tentare di risolvere, senza con questo voler disconoscere da parte nostra l'importanza fondamentale per l'agricoltura italiana dell'orizzonte europeo e del futuro della politica agricola comune. Come è già stato detto, gli obiettivi fissati nel 1958 durante la Conferenza di Stresa, e confermati dal Trattato di Lisbona, non sono stati raggiunti: il reddito degli agricoltori rimane ben al di sotto di quello medio complessivo ed è esposto a continue penalizzazioni dalla volatilità dei mercati. La bilancia commerciale dell'Unione europea è andata peggiorando, mentre il consumo del suolo avanza, nonostante gli infiniti richiami, a parole, alla multifunzionalità dell'agricoltura e al benessere che, oltre al cibo, può produrre per la collettività. Infine, c'è il cambiamento climatico: se 50 anni fa era difficilmente preventivabile, perlomeno nelle dimensioni assunte negli ultimi due decenni, fa piacere oggi per la condivisione della consapevolezza - vederlo richiamato nelle mozioni che guardano al futuro della nostra agricoltura, dopo che in questa stessa Aula abbiamo trascorso diverse ore ad ascoltare esponenti della maggioranza negarne la solidità scientifica, se non l'esistenza. Tant'è, pulpiti e predicatori si moltiplicano, mentre svaniscono idee e visioni che facciano presa sul reale. Ma torniamo alla nostra mozione e inizio, nel solco degli interventi che mi hanno preceduto, dagli impegni che il Gruppo dell'Italia dei Valori chiede al Governo a livello europeo. Le incongruenze, le iniquità e le inefficienze dell'attuale PAC vanno eliminate: la politica agricola comune non può ridursi a sostegno al reddito, ma deve essere l'occasione per la promozione di beni pubblici e di processi innovativi, in modo che il sistema agroalimentare possa diventare quel motore di sviluppo economico capace di gestire, con altri attori economici e sociali, il territorio rurale e le risorse naturali. A tal fine, il mantenimento dei *budget* della PAC va assicurato, perché gli agricoltori continuino a usufruire di benefici economici e sociali, ma vanno individuati criteri qualitativi di ripartizione, incentrati sul valore della produzione, anziché sull'estensione delle superfici. Così la PAC potrà essere un'autentica politica comune, senza distorsione della concorrenza, e sarà possibile garantire agli agricoltori un trattamento equo, tenendo conto della diversità di condizioni. Il ruolo degli agricoltori nella produzione economica va finalmente riconosciuto e rafforzato; a tal fine è indispensabile la tracciabilità dei prodotti, che garantisce la sicurezza alimentare a consumatori che, anche nella crisi, si rivelano sempre più consapevoli ed esigenti. Al contempo, la tracciabilità e un sistema di etichettatura che, nel quadro degli accordi commerciali, dia trasparenza alle indicazioni geografiche, possono assicurare competitività e un reddito equo agli agricoltori italiani ed europei: equo anche rispetto all'importanza della loro attività contro le sfide di questo terzo millennio, cioè il cambiamento climatico e la carenza di risorse idriche. una rete di sicurezza contro le crisi di mercato può essere rappresentata da un fondo anticrisi, basato su parametri e metodi di rilevazione comuni, è innegabile però che l'agricoltura italiana ha urgenza, ora, di scelte e risorse su cui, come ho già detto, il Gruppo dell'Italia dei Valori del Senato chiede al Governo impegni non più rinviabili. Ad esempio, abbiamo ormai indagini e dati sufficienti che testimoniano l'enorme divario tra il prezzo dei prodotti agricoli all'origine e quello al consumo. Il monitoraggio deve continuare, ma soprattutto sono indispensabili misure contro la speculazione. Così come, a fronte di una grande distribuzione che distorce il mercato e riempie i centri cittadini e le periferie di tir e rifiuti, è il consumo stagionale dei prodotti che va favorito, con incentivi alla filiera corta, spazi dedicati nei mercati e nei grandi magazzini, per aumentare le opportunità di offerta di prodotti locali e di qualità e ridurre il trasporto di merci su strada e il suo pesantissimo impatto ambientale. Le nostre imprese agroalimentari vanno sostenute, innanzitutto per il mantenimento dell'occupazione, al Sud in modo particolare, perché siano vitali sul fronte della ricerca e dell'innovazione, perché rappresentino un'opportunità per i giovani: in tal senso bisogna orientare le risorse, a partire dal rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, anche per la copertura del pregresso 2008-2009 e pervenendo ad una stabilizzazione triennale del Fondo stesso, alle agevolazioni contributive per le zone svantaggiate e ad interventi adeguati che consentano agli operatori zootecnici di far fronte alla grave crisi in cui versano. Concludendo, signora Presidente, onorevoli colleghi, vorrei invitare l'Aula a non sottovalutare l'occasione di riflessione e iniziativa che la discussione di queste mozioni ci offre, nonostante sia invalsa l'abitudine di considerare simili dibattiti un impegno che in pochi hanno a cuore, come si vede, per altri una recita dovuta, per molti un riempitivo

Qualsiasi tentativo di semplificare l'approccio alla politica agricola comune o di ridurne le variabili si scopre subito debole e inefficace, perché la complessità ci torna indietro come un boomerang. Che cosa fare allora per l'agricoltura italiana in Europa e nel mondo? Intanto cerchiamo di attribuire concretezza alle nostre parole, agli impegni che chiediamo e a quelli che ascolteremo dal Governo. È con questo invito, rivolto a tutti e a me stesso per primo, che mi dispongo all'avvio della pregando i colleghi da subito di non esercitare una memoria corta e settoriale: come ho già detto, parliamo di suolo, di acqua, di salute, oltre che di produzione agricola. Quel che diremo stasera in quest'Aula non potrà essere archiviato o cestinato, quando andremo a discutere di strade o di centrali nucleari, o di discariche e inceneritori. L'Italia questo è, signori:

del resto quella degli altri senatori che, con dovizia di particolari, hanno messo a fuoco le problematiche che riguardano il pianeta agricoltura. Io non ho lo stesso tempo a disposizione e quindi mi limito a soffermare l'attenzione sull'importante

fu sottoposto ad una sostanziale riforma che, con l'obiettivo di garantire la sopravvivenza degli ecosistemi senza per questo azzerare la competitività e la redditività del settore - avviò un processo di gestione a più lungo termine delle risorse ittiche: obiettivo, però, raggiunto solo in parte. Per questo motivo, adesso serve una riforma radicale della politica comune della pesca: una riforma che, sostenuta da stanziamenti di maggiore consistenza, favorisca uno sviluppo sostenibile del settore, in grado di assicurare elevati livelli di reddito e di occupazione per gli operatori e gli addetti; una riforma attenta alle ricadute sociali e ambientali degli interventi, rispettosa delle specificità regionali, soprattutto, più incentrata sulla pesca artigianale e costiera, che riguarda in modo particolare l'Italia. La nuova politica comune della pesca dovrà ispirarsi ai principi della regionalizzazione, della sussidiarietà e quindi tener conto delle caratteristiche specifiche dei mari europei. Sarà necessario adottare differenti modalità di gestione per la pesca d'altura e per quella costiera, assumere iniziative che incrementino la competitività dell'acquacoltura, attraverso un sostegno forte e continuo alla ricerca e allo sviluppo tecnologico del settore, rivolgere una particolare attenzione ai consumatori, assicurando un monitoraggio rigoroso, una tracciabilità completa dei prodotti immessi in commercio, anche e soprattutto di quelli provenienti dai Paesi terzi. E qui consentitemi una parentesi: non è concepibile che ancora non si riesca ad ottenere la tracciabilità, cioè l'etichettatura dei prodotti. Questo è molto grave perché l'Italia punta sulla qualità

Quindi bisogna assolutamente insistere in sede europea su questo problema, perché non è più tollerabile che prevalgano le *lobby* e i gruppi di pressione.

colleghi senatori, la mozione presentata dalla capogruppo del Partito Democratico in 9a Commissione, senatrice Pignedoli, ma anche molte delle altre discusse oggi in quest'Aula, evidenziano come la PAC futura rappresenti per il nostro Paese di fatto una riserva di straordinaria straordinaria opportunità di sviluppo. Era quindi importante portarla in discussione all'interno di quest'Assemblea perché si potesse anche noi, responsabili nella rappresentanza del nostro Paese, contribuire alla definizione della posizione dell'Italia. L'agricoltura e il sistema agroalimentare, nel suo complesso, si trovano oggi in una situazione inedita ed esclusiva di centralità nel sistema economico, sociale ma anche culturale del nostro Paese e di buona parte dei Paesi dell'Europa. La prima eccezionalità sta nell'intreccio tra le grandi sfide del nostro tempo e il ruolo di protagonista del settore primario: la sicurezza alimentare, l'emergenza cibo, la sostenibilità ambientale, la tutela del territorio e la stessa identità dei luoghi e delle comunità non possono essere risolti se l'agricoltura non ne sarà all'altezza. Il secondo elemento di eccezionalità risiede nella concomitanza tra la crisi strutturale del comparto, che si inserisce nella crisi economica più generale e più pesante dal dopoguerra, e l'ampio spettro di opportunità che oggi vengono offerte a questo settore. Non vi è nessun altro settore

il fatto che una parte di questi spinge per destinare parte del *budget* dell'agricoltura verso altri obiettivi di sviluppo rende sicuramente molto forte la competizione tra i Paesi. Per questo diventa importante che l'Italia sappia esprimere un piano strategico che dia prospettive nuove non solo al settore, ma all'intera economia dell'Europa, e su questo costruisca le proprie alleanze. Si tratta quindi di dire in modo chiaro qual è la strategia per la nuova politica comune: per noi è competitività e valorizzazione di quei beni pubblici che le imprese agricole sono in grado di produrre. Affrontare la sfida della competitività su produzioni di qualità e assumersi al contempo la responsabilità di garantire la produzione di beni pubblici, essenziali per le comunità, pone inevitabilmente al centro l'azienda e l'imprenditore agricolo, a cui la politica deve garantire un contesto favorevole e supportare

anche per superare una delle criticità più pericolose del settore, che solo se viene trasformata in elemento di forza può assicurare durata e respiro alle politiche. Il tema ovviamente è quello del ricambio generazionale. I dati sono sconfortanti in tutti i Paesi dell'Unione europea, ma in Italia sono peggiori. All'ultima rilevazione, gli imprenditori al di sotto dei quarant'anni, come abbiamo detto in tante occasioni, risultavano essere il 7 per cento, ma se guardiamo il parametro dei 35 anni, che è quello che definisce la

e dobbiamo farlo perché da qui di fatto arrivano i segnali più incoraggianti. Dai giovani imprenditori il messaggio è chiaro, forte e univoco, senza distinzioni, come dovrebbe essere univoca la voce che viene da quest'Aula:

politica agricola comune, questo ci chiedono i giovani imprenditori, questi credo che debbano essere anche i fondamenti della visione che il nostro Paese pone a fondamento della PAC; ed è questa

Invece una riflessione su questi argomenti è più che opportuna e necessaria: il settore primario è assolutamente importante, non solo per l'oggetto che tratta, non solo per il valore economico che ha nel complesso dell'economia nazionale, ma anche per l'immagine positiva e trainante che attraverso i prodotti di qualità dà un po' a tutto il nostro Paese ed anche per le nuove funzioni che l'agricoltura sta svolgendo. Penso alla tutela del paesaggio, alla gestione dell'ambiente, al turismo. È un dibattito importante, perché il settore è attraversato da una crisi profonda e diffusa: una crisi che continua, e che vede un calo degli scambi agroalimentari (si parla di meno 9 per cento per l'*import* e meno 11 per cento per l'*export*), perché c'è una volatilità dei prezzi eccessiva, perché sta calando il reddito delle imprese agricole, fino a porre molte di loro in una condizione di difficile sopravvivenza, e ancora, perché l'Europa, che pesa sempre più in questo settore, è alla vigilia di scelte importanti. La mozione che ho sottoscritto con i colleghi del PdL descrive bene questa situazione e indica con chiarezza al Governo gli obiettivi da perseguire; dunque mi limito ad alcune osservazioni più generali. La prima è la seguente. Non dimentichiamo che l'allargamento dell'Unione europea da 15 a 27 Stati, che ha comportato il passaggio del numero degli agricoltori da 6 a 13 milioni, l'aumento della superficie coltivata da 130 a 180 milioni di ettari e che vede tanta disparità nei livelli di reddito, se ha posto, pone e sicuramente porrà dei problemi, può essere anche una grande opportunità: pensiamo solo all'allargamento della platea dei cittadini consumatori, che arrivano a 500 milioni, e alla maggiore stabilità politica, dunque alla possibilità di programmare meglio e con più lungimiranza. è poi la PAC. La PAC si è rivelata uno strumento assolutamente valido anche per la nostra agricoltura. Dagli obiettivi iniziali, che erano, come è stato anche qui ricordato, quelli dell'incremento della produzione e del sostegno del reddito, la PAC ha saputo aggiornarsi, tenendo conto del cambiare della situazione e dell'agricoltura, ma anche più in generale dei cambiamenti avvenuti nella società. Adesso gli obiettivi cui tende, quelli della

Dunque, allargamento della Comunità europea positivo e PAC strumento valido, ma ad alcune condizioni, però, per l'avverarsi delle quali dobbiamo lavorare con la massima concordia possibile. La prima condizione è che l'ammontare globale dei finanziamenti dell'Europa per questo settore, o quantomeno quelli destinati al nostro Paese, non si debbono ridurre o ridurre troppo. L'Italia ha sempre avuto meno di quanto ha dato in questo settore e sarebbe inaccettabile per noi distribuire i fondi secondo il criterio della superficie, criterio sostenuto da alcuni Stati. Altra condizione è che poi questi finanziamenti che otteniamo li sappiamo sfruttare bene. Anche qui il nostro Paese ha sottovalutato storicamente il peso della Comunità ed è stato un errore che abbiamo pagato in diverse forme;

Al di là di questo, del rapporto con l'Europa e la PAC, ci sono delle scelte che dobbiamo compiere a livello di politica nazionale. Certo, anche in questi momenti di crisi finanziaria dobbiamo far sì che i fondi si riducano il meno possibile,

nuove. Ci sono troppi settori e troppi territori che vivono giorno per giorno secondo abitudini che non sono più consentite dalla normativa o dalla realtà economica che è mutata. Abbiamo un esempio che possiamo citare, assolutamente incontestabile e chiaro, di cosa non avremmo dovuto fare e di cosa non dobbiamo mai più fare rispetto a questi problemi. Mi riferisco alla vicenda delle quote latte.

- come ho già detto - richiedono un cambiamento di mentalità, ma anche una maggior collaborazione, un maggiore coordinamento fra i vari settori,

di saper interpretare la realtà, di parlare con chiarezza, di saper intrecciare rapporti positivi con gli altri colleghi, come dimostrano i contatti bilaterali che si sono tenuti in queste settimana a Roma. Ebbene, lo invitiamo a procedere in questo modo. Noi lo sosterremo con grande convinzione.

è evidente che le imprese agricole europee si confrontano oggi con una serie di sfide che impongono all'Unione europea scelte strategiche a lungo termine per l'avvenire. Non solo in agricoltura o nelle zone rurali, per assicurare adeguati livelli nella qualità della vita di tutti i cittadini. Sta per aprirsi la fase cruciale della negoziazione sulla riforma della politica agricola comune (PAC). La Commissione europea ufficializzerà infatti la propria proposta il prossimo 17 novembre e la nuova PAC dovrà entrare in vigore con il prossimo bilancio comunitario, quello del ciclo 2014-2020. Si tratta di una riforma epocale per la PAC

si deve sottolineare che in questi Paesi nuovi il settore agricolo è molto più esteso in rapporto all'economia rispetto all'Europa dei 15. Per avere un'idea delle proporzioni, basti pensare che il PIL dei Paesi del blocco orientale rappresenta meno del 10 per cento della UE a 25, mentre la loro superficie agricola è pari al 45 per cento dell'intera superficie agricola comunitaria e che, nonostante la produttività dell'agricoltura in questi Paesi è di gran lunga inferiore a quella media dei Paesi più avanzati, la loro produzione produzione agricola complessiva rappresenta circa il 30 per cento di quella totale della UE. È quindi un nuovo contesto quello a cui guardiamo, in cui ci troviamo ad operare e le questioni principali sul tavolo della riforma includono, in primo luogo, le dimensioni finanziarie della PAC nell'ambito del futuro bilancio UE; in secondo luogo, la riforma del sistema dei pagamenti previsti dalla PAC e, in particolare, il cosiddetto pagamento unico per azienda mirato al sostegno della produzione e dei redditi degli agricoltori e la eventuale introduzione di altre tipologie di pagamenti correlati ai beni pubblici ambientali da riconoscere solo agli agricoltori le cui attività producano effetti esterni positivi dal punto di vista ambientale. L'importanza del primo punto è evidente. Dato che è aumentato il numero di aziende e la dimensione complessiva del settore agricolo europeo, se l'ammontare delle risorse destinate destinate alla PAC non verrà aumentato o se addirittura venisse diminuito, ci saranno meno soldi per tutti in ogni caso e, quindi, meno soldi

degli stanziamenti del bilancio, per un ammontare complessivo che attualmente corrisponde a circa 50 miliardi di euro all'anno di erogazioni a favore degli imprenditori agricoli. Per quanto riguarda il secondo punto, anche qui si parla di risorse finanziarie che vanno ai Paesi membri. In particolare,

che a contendersi le risorse della PAC ora vi sono, a pieno titolo, anche gli agricoltori dei Paesi dell'Europa orientale da poco entrati nell'Unione europea. Le modalità di questa redistribuzione di risorse e, quindi, l'ammontare delle risorse PAC che i Paesi come l'Italia rischiano di perdere con la riforma dipenderanno proprio dal modo con cui sarà modificato il pagamento unico per azienda. Il terzo punto, anch'esso inerente la riforma del sistema dei pagamenti, è molto importante, perché è probabile che la Commissione europea ne faccia un punto qualificante della propria proposta di riforma.

sussidi diretti al sostegno della produzione e dei redditi delle aziende agricole e la loro sostituzione con erogazioni mirate a

cosa deriverebbe da questo? Il disegno di riforma che si va profilando trasformerebbe la PAC da strumento tradizionalmente dedicato al sostegno e alla garanzia dei redditi degli agricoltori europei a fronte della volatilità dei mercati e dell'erosione del valore aggiunto del settore agricolo, in un nuovo strumento Il peso dei due obiettivi nel disegno della nuova PAC dipende da quale delle due opzioni in campo si realizzerà e come peserà. Esistono diverse ipotesi di riforma: si va da un'ipotesi di semplice *upgrading* dell'attuale PAC che preveda solo pochi ritocchi al sistema attuale di pagamenti, all'ipotesi di una completa e radicale ristrutturazione della PAC. In questa seconda ipotesi si profilerebbe addirittura la soppressione

attiva e costruttiva e faccia sentire la propria voce. I punti su cui impegnarsi sono i seguenti: in primo luogo, puntare al mantenimento degli attuali stanziamenti per la PAC nell'attuale bilancio comunitario per fare in modo che siano sufficienti per le aziende di tutti i Paesi. In secondo luogo, il tavolo di riforma della PAC deve diventare l'occasione perché l'Italia ridisegni una propria politica economica per il settore agricolo: una nuova politica agricola nazionale con l'obiettivo di ridare slancio al settore agricolo italiano, non solo per consentirgli di mantenere e recuperare spazi nell'ambito del mercato agricolo europeo, ma per permettergli di conquistare nuovi spazi, anche nell'ambito extracomunitario, soprattutto attraverso la difesa del nostro *made in Italy* e delle nostre produzioni agroalimentari. Questo obiettivo richiede, certamente, che il settore recuperi la propria competitività, ma è imprescindibile che si eviti di penalizzare gli agricoltori italiani con una nuova PAC tutta sbilanciata a favore dei Paesi nuovi entranti nell'Unione europea e con una ripartizione delle risorse che tenga conto esclusivamente degli ettari di terreno agricolo e non valorizzi in modo opportuno

un minimo di certezza circa la continuità di remunerazione congrua, essi si trovano costretti in molti casi a chiudere le aziende, con conseguente progressivo abbandono di terreni e perdita di produzioni importanti per il nostro Paese. Le principali associazioni degli imprenditori agricoli hanno già lanciato l'allarme e manifestano difficoltà, in primo luogo, a causa della volatilità dei mercati agricoli e dei rischi derivanti dall'eccesso di produzione; in secondo luogo, a causa di un fenomeno che investe non solo il settore agricolo, ma che si estende a tutta la filiera agroalimentare: un fenomeno che vede l'aumento dei prezzi degli alimentari a valle per il consumatore finale accompagnato dalla riduzione delle remunerazioni a monte per gli agricoltori, a tutto vantaggio della fascia degli intermediari e della speculazione.

Signora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, la politica agricola dell'Unione europea è in continua evoluzione. Alle sue origini, cinquant'anni fa, la preoccupazione principale era garantire la produzione su vasta scala e l'acquisto delle eccedenze nell'interesse della sicurezza alimentare. L'attuale politica dell'Unione europea punta a far sì che i produttori di alimenti di ogni genere siano in grado di competere in modo autonomo sui mercati dell'Unione europea e su quelli mondiali. Il prossimo 17 novembre la Commissione europea dovrà presentare gli obiettivi e le linee strategiche della riforma della politica agricola comune *post* 2013. Nella strategia dell'Unione europea 2020, l'agricoltura e il sistema agroalimentare sono state inserite tra le sfide determinanti per contribuire ad una crescita dell'Europa verde sostenibile e per promuovere un'economia che assicuri alti livelli di occupazione e garantisca la coesione sociale e territoriale. La politica agricola europea ha subito una serie di importanti riforme negli ultimi anni. Il mondo agricolo in Italia paga purtroppo l'assenza di un'organica politica agraria nazionale. Non possiamo più rimandare una riforma della politica agraria nazionale con l'obiettivo di seguire un percorso più moderno per garantire la competitività delle imprese agricole. Infine, è necessario riorganizzare l'intero sistema primario. Il settore agricolo sta attraversando un periodo di grave e prolungata crisi. Dal 2000, mentre le imprese agricole europee sono cresciute in termini di competitività e redditività, quelle italiane sono rimaste al palo. Nell'ultimo anno il reddito agricolo è calato in Italia del 25,3 per cento, il doppio della media europea. I prezzi agricoli alla produzione hanno subito una flessione del 12,4 di conseguenza cresce l'indebitamento delle aziende. La progressiva riduzione della superficie agricola mostra una pericolosa tendenza all'abbandono e al degrado dell'ambiente rurale. Migliaia di agricoltori sono stati costretti a cessare l'attività agricola. Tra il 2000 e il 2007 l'agricoltura perde 474.000 aziende, un quinto del totale censito. Solo 112.000 aziende hanno una guida giovane. Nell'agricoltura italiana non vi è stato alcun ricambio generazionale. A tutto ciò vanno aggiunti i nodi non ancora sciolti, quali l'eccessiva frammentazione aziendale, gli alti costi di produzione e il peso della burocrazia. Non solo, la rapida e progressiva affermazione anche in Italia della grande distribuzione organizzata ha completamente modificato la modalità di distribuzione di prodotti agroalimentari e, allo stesso tempo, ha cambiato profondamente le relazioni tra i vari attori della filiera, imprese agricole comprese. Da ciò consegue che le prospettive della ripresa dell'agricoltura sono legate alla capacità di correggere il malfunzionamento dei mercati e di contrastare gli effetti della volontà dei mercati e delle manovre speculative. Per quanto riguarda la regolazione dei mercati, per esempio, vi è la necessità di organizzazioni economiche, nonché di accordi di filiera, e di una politica della concorrenza e della gestione dei rischi di mercato. Occorre in particolare rilanciare ed incentivare la commercializzazione sulla base di accordi contrattuali, introdurre più trasparenza nei processi di formazione dei prezzi prezzi lungo la filiera alimentare, garantire più informazione al consumatore a partire dall'etichettatura di origine, rafforzare gli strumenti di gestione dei rischi di mercato e i servizi finanziari finanziari volti a ripristinare i margini di liquidità delle imprese in situazione di crisi di mercato. Per aumentare la competitività delle imprese andrebbero stabilizzate alcune agevolazioni essenziali per la riduzione dei costi a carico delle imprese e previste due nuove misure finalizzate, la prima, a ridurre il costo del lavoro per le aziende operanti nelle zone ordinarie e, la seconda, ad estendere i benefici del credito d'imposta per gli investimenti a tutte le imprese agricole. Occorre poi semplificare il rapporto tra pubblica amministrazione e impresa agricola, realizzare il sistema di misurazione e controllo della burocrazia per indirizzare l'intervento del legislatore verso le aree di maggiore inefficienza, costruire l'anagrafe delle aziende agricole. Sarebbe inoltre opportuno definire un piano d'azione organico per sostenere il ricambio generazionale e incentivare la costituzione di nuove Le azioni da sviluppare per favorire l'attrattività e sostenibilità dell'attività agricola sono molte. Tra queste voglio ricordare la fiscalizzazione degli oneri sociali, misura cessata di recente, la reintroduzione del *bonus* gasolio, la stabilizzazione delle agevolazioni per l'acquisto dei terreni agricoli, la definitiva soluzione della questione ICI sui fabbricati rurali, le facilitazioni per gli imprenditori che investono in innovazione e ricerca. Sono queste le azioni da cui dovrebbe muovere il Governo nazionale sulla riforma fiscale per rilanciare l'agricoltura che sta attraversando una delle crisi più difficili degli ultimi 30 anni. I produttori fanno i conti con costi sempre più onerosi. I redditi, anche a causa del crollo dei prezzi sui campi, sono stati ridotti: solo lo scorso anno il taglio subito risulta superiore al 25 per cento, una situazione drammatica che impone immediati interventi. sotto il profilo fiscale, l'agricoltore non può pagare più di quanto già fa ora. Si richiedono inoltre alcune precise misure che alleggeriscano gli oneri burocratici per le imprese, mettendole in condizione di poter tornare a competere sui mercati. Consentitemi, a questo punto, di fare un cenno al futuro della politica agricola politica agricola comune nelle aree di montagna dopo il 2013. La tavola rotonda che si è tenuta a Bolzano lo scorso giugno ha evidenziato alcune realtà: il 40 per cento del territorio europeo è definito superficie agricola utilizzata; le aree svantaggiate di montagna occupano il 15 per cento di questa superficie, pari a 26,6 milioni di ettari e sono sparse in 16 Stati membri. L'Italia, dopo la Spagna, è il secondo Paese con la più vasta area montana; seguono Francia e Romania. Da soli, questi quattro Paesi rappresentano il 69 per cento delle aree svantaggiate di montagna dell'Unione europea. In alcune regioni appartenenti a questi Paesi, poi, il territorio è costituito al 100 da zone svantaggiate di montagna, queste regioni hanno, quindi, un notevole interesse a lavorare insieme per difendere la loro posizione e far valere i loro bisogni. Proprio a questo scopo, alcune regioni montane stanno lavorando insieme da alcuni anni: Trentino - Alto Adige, Friuli - Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Land Tirol, Freistaat Bayern, Land Vorarlberg hanno cominciato insieme un percorso nel 2008 ed ora vorrebbero coinvolgere altre regioni, con un'attenzione particolare a quelle spagnole. L'Unione europea in questi due anni pare aver compreso il valore delle zone di montagna e ha contribuito al loro mantenimento con specifici sostegni. Il futuro della loro agricoltura dipenderà molto dalle misure di intervento che l'Unione europea proporrà in seguito. *(Applausi

ritengo che i tempi risicati assegnati a questo dibattito siano lo specchio fedele del silenzio e dell'indifferenza con cui si guarda all'agricoltura del nostro Paese. Voglio solo ricordare ai presenti che esso riguarda la politica economica del Paese, che vale un fatturato di 220 miliardi di euro all'anno (il 15 per Tra l'altro, vedo anche un ritardo culturale, per il quale anche il mio partito porta delle responsabilità che, tuttavia, impallidiscono a fronte della delusione e dell'amarezza per quello che questo Governo

Ancora oggi, nella manovra di stabilità prevedete di tagliare quasi 220 milioni di euro. Ricordo a me stessa, poiché non avrò altre occasioni per poterlo fare, che questo avviene in una situazione che non è esagerato definire drammatica per l'agricoltura italiana: calo del reddito agricolo, che è il doppio di quello registrato nell'area UE; un progressivo invecchiamento degli addetti; un'ecatombe che ha visto chiudere tra il 2000 e il 2007 quasi mezzo milione di aziende agricole: non sono aziende travolte da criticità ed emergenze imprevedibili, lo dico a voi tutti. Siamo rassegnati al fatto che il Governo di cui lei fa parte non intende attuare per l'agricoltura quelle misure anticicliche cui hanno pensato Francia, Germania e così via: nessuna misura straordinaria, nessuna politica di sostegno. Cosa ancora più grave, non avete saputo - o, peggio, voluto - garantire agli agricoltori italiani la semplice ordinarietà, il quotidiano. Parlo, ad esempio, dell'odissea del rifinanziamento del fondo bieticolo-saccarifero, della proroga delle agevolazioni fiscali e contributive delle zone svantaggiate di montagna scaduto lo scorso 31 luglio o, ancora, del ripristino, eventualmente attraverso uno strumento alternativo, delle agevolazioni sul gasolio agricolo utilizzato per le coltivazioni sotto serra. Sono pochi esempi per i pochi minuti che mi sono concessi, ma lei sa, signor Sottosegretario, che potrei proseguire ancora a lungo. Ora viene in campo la discussione sulla riforma della PAC, la politica agricola comune, che noi del Partito Democratico abbiamo voluto discutere qui in quest'Aula. Come i colleghi sanno, è una partita che per l'Italia vale sei miliardi di euro e rappresenta l'occasione per ripensare un meccanismo ritagliato su misura per le grandi agricolture del Nord Europa, gravemente penalizzante per la varietà, la qualità e la tipicità delle colture mediterranee. Il Partito Democratico ha sottolineato, nella presentazione della mozione, che il pagamento unico paga l'estensione, ma non la qualità, la specificità e la varietà delle produzioni che, da sempre, sono il punto di forza del nostro *made in Italy*. Vanno, quindi, ripensati i termini dell'intervento pubblico, evolvendo da un intervento legato alla sola proprietà - ne parlava poc'anzi senatrice Poli Bortone - a meccanismi di premialità per comportamenti virtuosi e più coerenti con gli obiettivi della politica comunitaria. Dobbiamo cioè favorire chi crea lavoro; chi ha più capacità di impresa, di fare sistema, di creare maggiore efficienza di azienda, di accorciare le filiere; chi ha più capacità di innovazione e di prodotto; chi persegue la sostenibilità ambientale; chi ostacola fenomeni di rendita fondiaria; chi si impegna nei processi di trasparenza e informazione ai consumatori; chi lavora ai processi di nuova competitività dei mercati nazionali e internazionali basati sulla distintività e unicità del *made in Italy.* Percorsi che vanno incoraggiati, signor Sottosegretario, perché - mi rivolgo a tutto il Governo - le strade alternative sono quelle di cui abbiamo memoria in questi giorni: quelle fondate sui minori costi di produzione, quelle che vorrebbero spingere, come fa la FIAT di Marchionne, verso altre aziende, verso altri lidi. Via i diritti, più disoccupati, più povertà. Questo disegno iperliberista non ci interessa: noi non ci stiamo. Per questo, oggi siamo qui per discutere di politica agricola comune, ma anche di un pezzo della nostra politica economica. Tra gli obiettivi della nuova PAC, non possono non esserci anche politiche di sostegno al reddito dei produttori, anche e soprattutto per contrastare l'accresciuta volatilità dei prezzi, oltre qualità e salubrità del cibo secondo standard più elevati. A tale proposito, mi piacerebbe sapere come il Governo italiano intenda garantire la salubrità degli alimenti, non essendosi dotato, a differenza degli altri Paesi europei, di un *focal point* sulla sicurezza alimentare nazionale. Non so quante altre volte l'ho già detto in quest'Aula, ma voglio ricordare a tutti i colleghi senatori che in Italia, dove ci si preoccupa del falso *made in Italy*, dei falsi prosciutti e dei falsi formaggi, non esiste un *focal point* sulla sicurezza alimentare italiana. della politica agricola comune dobbiamo partecipare da protagonisti, per dare risposta alle imprese agricole, che sono oltre 1.700.000. Purtroppo, signor Sottosegretario,

i colleghi senatori) sulla base di quale confronto, di quale coinvolgimento il Ministro italiano delle politiche agricole va ad affrontare questa impegnativa scadenza. Ha parlato con qualcuno, ha chiesto il sostegno ed il supporto del Parlamento, ha ritenuto di confrontarsi con le organizzazioni agricole, con i sindacati, con le Regioni? Oppure andremo ancora una volta a ruota della Francia, della Germania e così via? Qual è la posizione italiana, del Governo italiano sulla politica agricola comune? Questo è quello che si chiede oggi in quest'Aula. Sono assolutamente persuasa e forse sono l'ultima rimasta in Italia (sottolineo l'ultima) - della solidità del Governo Berlusconi e della maggioranza che lo sostiene, ma, quando si tratta di rappresentare l'Italia in una sfida epocale, ogni contributo dovrebbe essere bene accetto. La sfida epocale di cui parlo, signor Sottosegretario, è quella di trasformare l'agricoltura in un'opportunità di lavoro per i più giovani, in un'occasione di sviluppo e di innovazione. Abbiamo tutti il preciso dovere di raccogliere la sfida, perché secondo me vi è un sodalizio indissolubile con la nostra storia, le nostre radici e la nostra identità. *(Applausi

Signora Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi senatori, gli obiettivi della politica agricola comune, fissati oltre 50 anni fa con la Conferenza di Stresa, sono stati recentemente confermati

ragionevoli per i consumatori. Purtroppo la recente evoluzione della politica agricola comune non ha consentito di cogliere tutti questi obiettivi, infatti: il reddito degli agricoltori rimane ben al di sotto di quello medio complessivo; la bilancia commerciale dell'Unione europea è andata peggiorando accumulando un pesante *deficit* commerciale; infine, i mercati sono tutt'altro che stabili ed espongono i redditi degli agricoltori a continue penalizzazioni; Tra l'altro, se effettivamente i consumatori hanno potuto godere di prezzi ragionevoli, ciò è accaduto a scapito della redditività dei produttori agricoli, che hanno avuto un ruolo sempre più subordinato nella filiera. Sarebbe necessario pertanto attuare una riforma della politica agricola comune che faccia perno sugli attuali strumenti (pagamenti diretti, misure di mercato e assi dello sviluppo rurale), secondo una nuova articolazione che abbia per obiettivo la semplificazione degli strumenti e delle procedure, la finalizzazione degli interventi a favore degli agricoltori professionali, la valorizzazione del ruolo del settore agricolo per la crescita economica e l'occupazione, la qualificazione dell'attività agricola per fronteggiare adeguatamente le sfide globali; il tutto operando «gradatamente gli opportuni adattamenti» come previsto dal Trattato. In ogni caso, prima della fissazione delle prospettive finanziarie per il 2014-2020, andrebbero opportunamente definiti i principi, i criteri direttivi ed i fabbisogni della riforma della politica agricola per i prossimi anni. Sinora i pagamenti disaccoppiati sono stati erogati ai beneficiari storici perché compensativi di una situazione pregressa, poi venuta meno, che concedeva agli agricoltori determinate garanzie di prezzo e di mercato. Oggi, questa voce di spesa rimane comunque determinante per il reddito degli agricoltori e, conseguentemente, per i beni pubblici che il settore agricolo garantisce alla collettività. Ciononostante, il criterio di assegnazione su base storica dei pagamenti diretti disaccoppiati non risulta del tutto giustificabile dopo diversi anni di applicazione. Esso, inoltre, sta rischiando di generare disparità di trattamento tra soggetti beneficiari e comparti produttivi. Si ritiene pertanto possibile avviare la discussione sul superamento del criterio della storicità, riformando, ad esempio, l'attuale sistema in primo luogo attraverso un pagamento di base ad ettaro destinato a compensare il carattere particolare dell'attività agricola, calcolato utilizzando come riferimento l'attuale massimale finanziario dei pagamenti diretti di ciascun Paese. Tale pagamento rimarrebbe assoggettato alla condizionalità, esclusivamente alle misure obbligatorie oggi già previste dalla normativa, eliminando invece tutti i requisiti stabiliti oltre le prescrizioni obbligatorie di legge. In secondo luogo, si potrebbe prevedere un pagamento aggiuntivo ad ettaro, commisurato in base a parametri oggettivi fissati forfetariamente a livello di Stato membro e correlati a due categorie di fattori. dalla situazione strutturale oggettiva in cui opera l'azienda agricola e dai comportamenti tesi alla salvaguardia ambientale. In particolare, utilizzando l'ammontare finanziario attualmente destinato a tale scopo nell'ambito dello sviluppo rurale, si potrebbe assegnare un importo di riferimento aziendale

concesso in base alla necessità di rispettare la normativa comunitaria che va al di là degli standard internazionali; all'adozione di comportamenti in linea con l'esigenza di fronteggiare

Presidente, onorevoli colleghi, con chiarezza è emersa dal dibattito una condivisione, già leggibile nel testo delle mozioni, su quelle che dovrebbero essere le linee guida del Governo in vista della riforma della PAC. senz'altro patrimonio comune questo potenziale ruolo multifunzionale dell'agricoltura, a partire dalla fondamentale produzione di cibo: salvaguardia del territorio e delle sue tradizioni, tutela della biodiversità e delle risorse idriche. una ricchezza potenziale che va salvaguardata, anche grazie al mantenimento del *budget* europeo destinato all'agricoltura. Vanno però modificati - e anche in questo caso si tratta di un obiettivo condiviso - i criteri di attribuzione delle risorse: superamento delle serie storiche, valorizzazione delle differenze, quindi delle eccellenze e delle produzioni che assicurano qualità ambientale e sociale. Tutto questo avrà un senso se sarà garantita anche la trasparenza delle importazioni in Europa, per la corretta informazione dei consumatori e la tutela del reddito e della qualità della vita degli agricoltori italiani ed europei. Insomma, al Governo italiano abbiamo chiesto di considerare l'agricoltura, sul tavolo europeo della riforma della PAC, un motore indispensabile della *green economy*. Tornando a quell'invito al senso di concretezza che ho rivolto all'Aula illustrando la mozione dell'Italia dei Valori, non posso in questa sede evitare di confrontarmi con i testi proposti dai Gruppi di maggioranza, di cui ho già comunque indicato gli aspetti di condivisione. Ad esempio, i colleghi senatori della Lega sembrano preoccupati da una sorta di competizione, in termini di accaparramento di porzioni di territorio, che può determinarsi tra produzioni di energia da fonti rinnovabili - quali l'eolico e il solare - e l'agricoltura, che meglio sarebbe salvaguardata dando priorità a fonti rinnovabili di origine agricola. Attenzione però, perché il discorso è fondato e, al tempo stesso, insensato: il consumo delle aree agricole la desertificazione del suolo in Italia si sono determinati per l'assenza di programmazione e per una frenesia di sviluppo concentrata solo sull'appagamento di appetiti immediati: soldi e consenso facili. Col precipitare della crisi economica, di questo sviluppo ci sono rimasti dissesto idrogeologico, aree abbandonate e cemento sul letto dei fiumi. La produzione di energia, cari colleghi, va programmata, è oggetto di scelte e di decisioni: servono il piano energetico nazionale e piani energetici regionali. O forse pensate che fonti rinnovabili di origine agricola non possano poi diventare competitive esse stesse con produzioni agricole destinate all'alimentazione e al mercato? O pensate che gli agricoltori che si trovassero a lavorare non lontano da una centrale nucleare potrebbero ricavare vantaggi competitivi dalla "tracciabilità" dei loro prodotti? Non si tratta di inventarci ulteriori motivi per dividere un popolo già drammaticamente frammentato nella difesa di piccoli e grandi interessi, e spremere consenso territoriale. Conoscenza, scelta e programmazione per la collettività e le generazioni di oggi e di domani: a questo è chiamata la politica. al Governo ed alla maggioranza l'urlo di dolore del ministro Galan, il quale, dopo il Consiglio dei ministri che ha licenziato il disegno di legge di stabilità ora all'esame della Camera, Non ci sono soldi, non c'è programmazione - chissà che cosa pensa il ministro Tremonti dei nostri sforzi di ragionare oggi sulla riforma della PAC del 2013! - e gli errori sono numerosi. Nella mozione, signor Sottosegretario, abbiamo voluto citare una vicenda emblematica: la vendita, da parte del gruppo Conserve Italia, del marchio De Rica alla multinazionale Olam International, che lo potrà utilizzare per commercializzare prodotti in Africa e nei Paesi dell'emisfero australe. Una finanziaria pubblica, con socio unico il Ministero delle politiche agricole, ha dato un consistente aiuto a questa operazione, che ha contribuito a sradicare un'attività tipica del Mezzogiorno per trasferirla dapprima al Nord, e vendere poi un marchio famoso in Italia e nel mondo ad una multinazionale che lo trasferirà in Africa,

avuto modo di dire in precedenza. Signor Presidente, non potevo sottolineare quanto condividiamo e tacere su discrasie, errori e contraddizioni senza venir meno a quell'impegno di concretezza che dall'inizio ho chiesto all'Aula e a me stesso.

Sottosegretario, la discussione, per quanto indubbiamente breve, mi è sembrata seria ed approfondita, così come deve essere quando si ha la responsabilità di affidare ad un Ministro l'onere di sostenere in sede comunitaria Abbiamo analizzato le conseguenze anche negative dell'attuazione della PAC, la sua evoluzione nel tempo, l'aggiunta di un secondo pilastro che tanto influisce sul riorientamento complessivo della politica comune. Mi pare che le riflessioni che ci uniscono siano più di quelle che ci dividono. infatti, parlato solo del pur necessario mantenimento del *budget*, ma soprattutto del valore del lavoro agricolo, che deve essere tutelato come bene prezioso della nostra Nazione: tutelato, difeso, accompagnato, incentivato nell'aspirazione di coniugare tradizione e modernità, identità e mercato, ambiente, produttività, reddito. È una sfida non da poco, che presuppone risposte ambiziose quanto precise e puntuali. Mi pare che il nodo centrale della riforma, cioè il futuro del sistema di pagamento disaccoppiato, sia stato trattato con notevoli affinità di valutazione. Non possiamo accettare che la redistribuzione del *plafond* degli aiuti diretti fra i 27 Stati membri penalizzi l'Italia, che, come abbiamo visto, ha dalla sua un notevole valore della produzione dovuto a più fattori. Dobbiamo evitare, quindi, in sede europea che la Commissione insista sul considerare il valore della produzione una sorta di variabile indipendente, ininfluente rispetto al considerare la superficie agricola quale unico parametro per la redistribuzione degli aiuti. È un forte elemento di criticità che va superato, anche in considerazione della valorizzazione del secondo pilastro

agricoltura-ambiente, che meglio potrebbe rispondere alle esigenze della PAC, senza per questo impoverire ulteriormente le risorse squisitamente del settore agricolo. Non è la superficie che può fare la differenza, ma la qualità e la quantità del lavoro, le capacità imprenditoriali e di innovazione, il saper rispondere adeguatamente all'evoluzione della domanda dei consumatori europei. Bisognerà, in Europa, saper dare sostanza a quel grande interesse che ha l'Italia di rendere più leggibile e forte e il rapporto fra sostegno e produzione di beni pubblici, intendendo per tali tutti i prodotti identitari legati al territorio, la salubrità, la qualità degli alimenti, la sicurezza alimentare, l'agricoltura sociale, il paesaggio, la valorizzazione diversificata dello spazio rurale. Sarà importante sostenere il pur previsto sistema di consulenza aziendale in modo che gli agricoltori siano realmente informati sull'evoluzione dei processi aziendali. Perché non pensare anche ad eventuali supporti tecnici a disposizione di quelle fasce più deboli di agricoltori poco avvezzi ad avvicinarsi, ad esempio, ai temi della ricerca e dell'innovazione? La PAC, insomma, proprio per essere una politica comune europea, deve avere degli obiettivi che siano realmente ambiziosi. Se vogliamo che l'agricoltura riprenda la sua vivacità dobbiamo agevolare gli incentivi collegati ai risultati ed alleviare gli agricoltori dai pesanti costi di produzione che oggi subiscono, nonché dalla pressione fiscale sul loro redditi, che è diventata tanto insopportabile da essere una delle cause prime dell'abbandono e della trasformazione dell'agricoltore in una sorta di "affittasuoli" per impianti energetici, con tutti i danni evidenti sia per l'impoverimento del settore primario che per la devastazione delle identità territoriali. È utile fare Come sosteneva con puntualità il collega Pinzger, per essere forti in Europa nella richiesta, dobbiamo noi avere in Italia un'organica politica agraria nazionale. È un dibattito, signor Sottosegretario, che da qualche tempo stiamo chiedendo a gran voce, una politica che in primo luogo faccia sì che le disuguaglianze che vogliamo eliminare in Europa non ci siano più in Italia; che gli agricoltori italiani tutti, sia che operino in zone svantaggiate o in zone di montagna, al Nord come al Sud, possano crescere in termini di redditività e competitività al pari di una qualsiasi impresa agricola europea. In Italia l'agricoltore sta soffrendo. Nella crisi generale forse soffre più degli altri: prezzi agricoli giù, reddito giù, costo del lavoro esoso, mancanza d'informazione, assenza di di consulenza organizzata, mancato ricambio generazionale, costi di acqua e di energia, carenze ed incapacità di alcune Regioni, persino di mettere a frutto le risorse comunitarie. Nella Decisione di finanza pubblica recentemente approvata abbiamo ottenuto l'impegno del Governo ad intervenire per la fiscalità di vantaggio, il credito di imposta per le aziende (naturalmente, comprese quelle agricole), la priorità per le infrastrutture (perché anche la carenza di trasporti idonei genera una forte aggravio di costi, e quindi una minore competitività). Tutte cose che conosciamo - tutti noi - e che credo ciascuno vorrebbe poter sapere affrontare e risolvere. Mi piacerebbe, ci piacerebbe, in prossimità dell'appuntamento europeo, signor Sottosegretario, che l'Italia andasse non solo con le idee chiare, ma con una voce - lo ribadisco ancora una volta - unica e forte, rimandando il dibattito franco e leale sulla politica agricola nazionale ad altro momento, pur necessario ed urgente. In Italia, sappiamo tutti che ci sono problemi insoluti. C'è ancora assenza di misure anticicliche; ci sono tagli in sede di bilancio nazionale, che non sono giustificabili nemmeno in una situazione riconosciuta di crisi. Allora, noi chiediamo di evitare di privilegiare alcuni e di danneggiare altri. Lo chiediamo in Europa, ma allo stesso modo chiediamo al Governo italiano di non soffocare il settore primario, ma di conferirgli in Italia quella dignità

che si possa realmente discutere della nostra politica nazionale. Non è vero infatti che gli interventi non si possono fare; tutto sta a saper scegliere le priorità. Io ritengo che l'agricoltura italiana abbia ancora il merito di aver saputo mantenere non soltanto la dignità del settore primario, ma anche l'economia della nostra Italia, oltre che quella tutela dell'ambiente alla quale abbiamo tenuto prima ancora che l'Europa ce la indicasse come obiettivo.

Signor Presidente, egregi colleghi, signor Sottosegretario, la mozione presentata dal Gruppo Lega Nord ha l'evidente scopo di sensibilizzare il Governo in vista dell'appuntamento sulla riforma della politica agricola comune. La nostra agricoltura sta scontando evidenti difficoltà di adeguamento al nuovo contesto delineatosi a seguito delle quattro successive riforme che, in meno di vent'anni, hanno pressoché stravolto l'originario assetto della originaria politica comunitaria.

debba chiaramente essere competitiva, e quindi debba far ottenere ai nostri agricoltori dei redditi remunerativi, che oggi non sono tali, in un mercato ormai aperto ad una competizione che non si ferma più al contesto europeo, ma è sicuramente su scala mondiale. In passato, non sempre è stata posta adeguata attenzione all'evoluzione del quadro comunitario ed internazionale, e quindi alla necessità di adeguare il nostro sistema produttivo agricolo ai nuovi scenari che, a seguito di tali evoluzioni, si sono delineati nel tempo. Purtroppo, lo scarso impegno del passato, che annovera tra i tristi risultati anche la trista vicenda delle quote latte, non deve assolutamente ripetersi in futuro. Adesso siamo nell'imminenza di una nuova fase di adeguamento che attende la PAC e che condurrà alla definizione di ancora nuovi assetti per il prossimo periodo di programmazione finanziaria, che inizierà nel 2013 e andrà ad ultimarsi nell'anno 2020. nell'anno 2020. Questa nuova prospettiva di adeguamento dei contenuti della PAC, giova evidenziarlo, pone problemi di assoluta importanza, come la quota di risorse che, sul totale del bilancio comunitario, dovranno essere destinate all'agricoltura, il miglioramento dei meccanismi di distribuzione del sostegno, sia tra gli agricoltori, sia tra i due pilastri in cui continuerà ad essere articolata la stessa PAC. In questa importante PAC. In questa importante prospettiva, occorre maturare piena consapevolezza che dalla PAC sicuramente discenderanno i principali strumenti per assicurare il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole nei nostri territori. A questo riguardo ci sembra che, non solo a livello comunitario ma, talvolta, anche in Italia, si stenti a maturare una piena consapevolezza riguardo all'effettiva importanza sociale ed economica che investe la presenza delle attività produttive agricole nel nostro territorio e, quindi, alle conseguenze negative a cui sarebbe esposto il nostro intero sistema socioeconomico nell'eventualità di un drastico ridimensionamento del nostro sistema produttivo agricolo. Il nostro territorio nazionale è costituito per il 76,8 per cento da aree collinari e montane e per più dell'80 per cento da aree rurali, dove l'agricoltura, anche quando non è in grado di svolgere un ruolo economicamente decisivo, contribuisce, comunque, notevolmente a determinare le caratteristiche sociali, ambientali e paesaggistiche.

oggi ad essere fondato su piccole comunità e piccole imprese, le cui possibilità di sviluppo sono indissolubilmente legate al contesto territoriale e agricolo. In questo senso, occorre avere chiaro che, in una prospettiva come quella attuale, la gran parte dei sistemi socioeconomici presenti a livello territoriale è evidentemente esposta al rischio del sottosviluppo e della marginalizzazione, qualora la politica non sia in grado di dare ulteriori possibilità oltre a quella di doversi misurare sugli standard di competitività imposti dalla crescente apertura dei mercati. La nostra agricoltura, per la grande complessità ambientale e sociale che la caratterizza, non può unicamente legare il proprio futuro alle fragili suggestioni del libero mercato, ma deve impegnarsi a scoprire autonomi percorsi di sviluppo fondati sulla valorizzazione delle proprie risorse umane, ambientali e produttive. È assolutamente necessario un preciso progetto politico in grado di tutelare e migliorare le diverse identità della nostra agricoltura e di costruire, per ciascuna di esse, una dimensione propria nell'ambito dello spazio globale che va definendosi a livello planetario. Diversamente, si rischia di mettere a repentaglio la sopravvivenza di quello straordinario patrimonio ambientale, economico e culturale che è costituito dai rapporti che legano l'agricoltura al territorio, alla natura ed alla società. Noi della Lega Nord auspichiamo un'agricoltura più redditizia, più efficiente nell'uso delle risorse, con maggiore attenzione e sensibilità agli aspetti ambientali, maggiore trasparenza e valorizzazione della qualità e della salubrità dei prodotti messi sul mercato. Personalmente, mi dispiace di dover contraddire il collega Di Nardo quando parlava di particolare preoccupazione della Lega Nord su temi che invece noi intendiamo supportare: mi riferisco al fotovoltaico. Noi non vogliamo utilizzare il terreno agricolo e sfruttarlo allo scopo di produrre reddito con il fotovoltaico, ma riteniamo che i tetti delle aziende possano sicuramente essere utili per portare un valore aggiunto alla redditività dell'impresa. dell'impresa. Riteniamo di dover valorizzare ed esaltare la grande potenzialità che ci viene dalla biodiversità di cui la nostra agricoltura è ricca. Siamo i primi produttori europei di prodotti biologici; possiamo vantarci di ben 4.396 specialità alimentari tipiche censite ufficialmente dalle nostre Regioni; abbiamo ben 177 tra prodotti DOP e IGP; deteniamo da soli ben il 22 per cento dei prodotti certificati in Europa. L'intervento pubblico a sostegno dell'agricoltura, se escludiamo le agevolazioni fiscali e contributive, è oramai quasi integralmente determinato dai finanziamenti di fonte comunitaria attraverso i piani di sviluppo regionali. Ne discende che non possiamo più permetterci di osservare distrattamente le evoluzioni del quadro comunitario, ma che dobbiamo impegnarci affinché la nuova PAC sia coerente con gli interessi e le potenzialità di sviluppo della nostra agricoltura. Dobbiamo contribuire attivamente alla costruzione della nuova PAC, non subirla passivamente come è successo per il passato. Per questo, riteniamo sia importante e doveroso impegnare il Governo ad adottare tutte le iniziative necessarie, affinché la nuova fase di revisione della PAC sia vissuta da protagonisti, partecipando attivamente alla definizione dei nuovi interventi, e, in particolare, a fare in modo che non vi sia un ridimensionamento dell'impegno comunitario in favore dell'agricoltura. I nuovi strumenti comunitari debbano essere definiti nel rispetto delle caratteristiche dell'agricoltura stessa in specie, del suo ruolo territoriale e della complessità dei rapporti che la legano alle altre componenti del nostro sistema socioeconomico. Tutto questo, chiaramente, a supporto del reddito dei nostri agricoltori e delle attività delle aziende agricole.

i nostri saluti e gli auguri per la loro attività di studio. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di voto ricordando - e mi riallaccio all'intervento fatto prima in discussione generale - che gli obiettivi della politica agricola comune prevedono l'incremento della produttività, il miglioramento del reddito degli agricoltori, la sicurezza degli approvvigionamenti, la stabilizzazione dei mercati e prezzi ragionevoli per i consumatori. Dobbiamo anche ricordare, votando queste mozioni, che il reddito degli agricoltori rimane ben al di sotto di quello medio complessivo. La bilancia commerciale dell'Unione europea è andata peggiorando, accumulando un pesante deficit commerciale, e i mercati sono tutt'altro che stabili ed espongono i redditi degli agricoltori a continue penalizzazioni. Tra l'altro, se effettivamente i consumatori hanno potuto godere di prezzi ragionevoli, ciò è accaduto a scapito della redditività dei produttori agricoli, che hanno avuto un ruolo sempre più subordinato nella filiera. Pensiamo allora ad una riforma secondo una nuova articolazione, che abbia per obiettivo, per esempio, la semplificazione degli strumenti e delle procedure, la finalizzazione degli interventi a favore degli agricoltori professionali, la valorizzazione del ruolo del settore agricolo per la crescita economica e per l'occupazione, la qualificazione dell'attività agricola per fronteggiare adeguatamente sfide globali che continuamente si propongono: il tutto, operando gradatamente gli opportuni adattamenti, come previsto dal Trattato. dal Trattato. Quindi, nel dichiarare il voto favorevole del Gruppo Futuro e Libertà per l'Italia alla mozione sottoscritta, quale secondo firmatario, dal senatore Digilio, capogruppo in Commissione agricoltura del Gruppo Futuro e Libertà, voglio ricordare che la stessa contiene quei punti che già ho sottolineato nel corso della discussione generale e che credo siano importanti, come la partecipazione attiva all'elaborazione della riforma della PAC, il mantenimento dell'attuale livello di finanziamento della PAC nell'ambito del bilancio comunitario,

con riferimento agli interventi di gestione del mercato per fronteggiare la volatilità dei prezzi, uno dei punti fondamentali e dei pericoli maggiori), la previsione di misure specifiche per favorire l'accesso diretto degli agricoltori al mercato, la revisione del pagamento unico aziendale, il miglioramento della trasparenza del mercato e la garanzia a livello europeo che le importazioni rispettino le norme comunitarie in materia di sicurezza alimentare. Nel

che il Parlamento non si trovi più a dover approvare emendamenti come quello sulle quote latte, che è stato, a nostro giudizio, uno schiaffo in faccia ai tanti produttori di latte che si sono sempre comportati onestamente ed hanno sempre provveduto regolarmente ai loro pagamenti. *(Applausi

*(PD)*. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, l'iniziativa che il Gruppo del PD in Commissione agricoltura ha assunto sotto la guida del Capogruppo, senatrice Leana Pignedoli, depositando, in data 4 agosto, una mozione sulla politica agricola comune, rappresenta un gesto di grande responsabilità. Ci siamo determinati a compierlo dopo aver registrato l'assoluta stagnazione del dibattito su un tema così importante e la mancanza d'iniziativa da parte del Governo. Sarebbe stato legittimo attendersi l'attivazione di tavoli di confronto con il mondo professionale, con le sue organizzazioni, con la cooperazione, i sindacati, con le Commissioni agricoltura in entrambi i rami del Parlamento, con il Presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, che è un italiano - non dimentichiamolo - l'onorevole Paolo De Castro, già senatore e prima ancora più volte Ministro per le politiche agricole, e naturalmente con le Regioni. È indubitabile l'utilità di un approfondimento su un tema così importante e di una conseguente posizione italiana in merito. Va detto che il commissario europeo all'agricoltura, Dacian Ciolos, promosse una consultazione pubblica sulla PAC che ha stimolato attenzioni ed interessi sull'intero territorio dell'Unione europea, trovando assente, quanto meno sul piano dell'iniziativa pubblica, il Governo italiano. Del resto, a me pare che tale atteggiamento sia in linea con le reiterate disattenzioni del Governo nei confronti dell'agricoltura, che ancora e per l'ennesima volta il Gruppo del PD in quest'Aula ha variamente stigmatizzato durante il recentissimo dibattito sulla Decisione di finanza pubblica, e che hanno trovato, ahimè, puntuale riconferma nella legge finanziaria approvata di recente in Consiglio dei ministri, tanto da suscitare la reazione dello stesso titolare delle Politiche agricole, onorevole Giancarlo Galan, che avremmo voluto quest'oggi presente in Aula, come ha giustamente rilevato la collega Mongiello (non se ne dolga il sottosegretario Buonfiglio, perché nulla è sottratto alla sua autorevolezza). Era indispensabile costruire una posizione nazionale in vista della riforma della politica agricola comune, a partire dalle acquisizioni che, in un tempo non lontano, esattamente a fine 2008, a proposito della verifica di medio termine, il cosiddetto *health* *check* della PAC, portarono in evidenza l'argomento. Il Partito Democratico in quella fase - come ha fatto nuovamente ai primi di settembre di quest'anno nell'ambito della festa nazionale del PD per l'agricoltura a Reggio Emilia invitò il relatore in Parlamento europeo, onorevole Capoulas Santos, offrendo così l'opportunità anche a parlamentari della maggioranza e alle rappresentanze del mondo agricolo di trarre spunti e di attingere informazioni da fonte particolarmente autorevole e competente.

fissare obiettivi condivisi in modo che si possa recuperare terreno e, nei successivi passaggi, come quello nodale del Consiglio dei ministri agricoli dell'UE, l'Italia possa esibire una posizione che rappresenti veramente la migliore sintesi la migliore sintesi delle più avvertire necessità del settore e indicare le modalità attraverso cui offrire risposte con gli strumenti di cui la PAC può ragionevolmente disporre; ciò anche in considerazione della penuria di risorse nazionali e dei tagli ripetuti alle voci di spesa per il comparto agricolo. È evidente che andranno assunte iniziative e stipulate alleanze con Governi di altri Paesi in modo da scongiurare, come è ben chiaro, pericoli di marginalizzazione o addirittura di isolamento dell'Italia. I problemi che abbiamo dinanzi sono in primo luogo relativi allo stanziamento di bilancio europeo per la spesa agricola, tenendo oggettivamente conto della spinta che pur proviene dai 12 Paesi di più recente adesione all'Unione. L'impegno deve tendere sempre più all'obiettivo della conferma dell'attuale stanziamento. Con riferimento poi al merito, la riforma deve incentrarsi sugli attuali strumenti (pagamenti diretti, misure di mercato e assi dello sviluppo rurale), secondo una nuova articolazione che miri alla semplificazione delle procedure, alla finalizzazione degli interventi a favore degli agricoltori professionali, alla valorizzazione del ruolo del settore agricolo per la crescita economica e l'occupazione e quale insostituibile strumento di salvaguardia ambientale, alla qualificazione dell'attività agricola per fronteggiare adeguatamente le sfide globali, all'innovazione tecnologica e al sostegno all'imprenditorialità femminile e giovanile. Sullo sfondo di questo scenario vi è sempre la finalità - che non possiamo rinunciare a raggiungere, malgrado la negligenza del Governo - di una vera e propria politica agricola nazionale, capace di riprendere il passo e di stabilizzare il reddito agricolo grazie all'intervento europeo. Ciò corrisponde all'auspicio che al più presto il Governo italiano si accorga che anche dall'agricoltura possono trarsi risposte efficaci alla crisi economico-finanziaria e alla disoccupazione. Le azioni per lo sviluppo rurale previste dalla PAC dovranno sostenere gli investimenti, incoraggiare il ricambio generazionale, recuperare in competitività, favorire l'integrazione di filiera e la promozione dell'*export*. Recentemente, a Lecce, in occasione dell'annuale conferenza economica della CIA, cui ha partecipato il Ministro per le politiche agricole (ed era presente tra i relatori anche il presidente della Commissione agricoltura del Senato, del Senato, Scarpa Bonazza Buora), è stato presentato un documento congiunto della medesima Confederazione italiana agricoltori, di Confagricoltura e di Copagri, che contiene alcuni spunti interessanti e per larga parte condivisibili in quanto estremamente oggettivi. La mozione del Partito Democratico ritorna sulla necessità di garantire un momento di confronto adeguato non soltanto con le organizzazioni professionali,

del Partito Democratico, dai colleghi della maggioranza che siedono in Commissione agricoltura e dalle altre mozioni sull'argomento, rappresenti un patrimonio da non disperdere, sul quale anzi fondare il presupposto per dare risposte vere al comparto agricolo. Il Gruppo al quale mi onoro di appartenere insiste da due anni e mezzo

che hanno presentato mozioni e tutti i colleghi intervenuti oggi abbiano conferito al dibattito che da tempo si sta svolgendo nel nostro Paese in materia di politica agricola comune un particolare rilievo.

a parlare di politica agricola comune, ci sarebbe il pienone, non basterebbero tutte le balconate che sono attorno a noi e sarebbero presenti tutte le televisioni. Questo, in Italia non avviene, anche se tutti sappiamo - e molti colleghi lo hanno ricordato - che abbiamo la seconda agricoltura d'Europa

una posizione italiana che deve essere interpretata nel modo più autorevole da parte del nostro Ministro dell'agricoltura. Quindi ci disporremo di conseguenza, signor Presidente.

siamo passati a tappe forzate e forse troppo veloci a riforme continue. Anch'io sono un riformista: chi non è riformista nel nostro Paese è un perdente, e io preferisco stare con i vincenti, e inoltre è giusto essere riformisti. Tuttavia troppe riforme

anche come agricoltore, visto che sono orgoglioso di esserlo. *(Applausi dal Gruppo PdL).* Dobbiamo puntare alla conferma del *budget* comunitario per l'agricoltura:

eccellenza Sottosegretario - come si diceva una volta - colleghiamoci alla linea francese o tedesca, nella consapevolezza che quella inglese è molto distante dalla nostra,

alla Camera dei deputati - qualcosa che sia funzionale al nostro interesse specifico. Vado rapidamente a concludere. Una volta conseguito il *budget* comunitario e conseguito il *budget*

Vanno riservate a chi fa effettivamente agricoltura imprenditoriale e professionale, e da questo punto di vista noi abbiamo già un parametro di riferimento, che è quello che fu stabilito dal decreto legislativo n. 99 del 2004 - dell'allora ministro Alemanno e del sottoscritto, suo Sottosegretario

di imprenditori agricoli e non agricoli che si costituiscono in società agricola e danno luogo ad un'entità imprenditoriale professionalmente riconosciuta. Questo è fondamentale

bensì un Presidente del Consiglio molto impegnato, un Ministro dell'economia che porterà a casa un *budget* agricolo importante, un Ministro dell'agricoltura che con grande umiltà,

di spadone tra di noi, oggi è giornata per chiarirci le idee tra di noi e consegnare al ministro Galan una proposta che sarà la sommatoria di tutto quello che è stato detto oggi, che sicuramente gli servirà

gli impegni che noi vorremo fargli prendere come suo Gruppo di riferimento, ma anche, credo, i consigli, assolutamente intelligenti ed amichevoli, che gli vengono rivolti da importanti Gruppi dell'opposizione.

presente in tribuna una rappresentanza del Consiglio comunale di Stimigliano, in provincia di Rieti,

le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

Se ci sono quelli che votano a favore e quelli che non partecipano al voto, secondo voi qual è la valutazione? Volete venire voi qui e decidere qual è il risultato? Informatevi e seguite il dibattito.

le agenzie hanno battuto la notizia della condanna a morte per impiccagione di Tareq Aziz. È in corso una mobilitazione internazionale; il Governo italiano ha già fatto sentire la propria voce, come anche

una scelta giusta, visto che il nostro Paese è contro la pena di morte e si è impegnato all'ONU affinché venisse decisa una moratoria. Anche l'Unione europea è dello stesso avviso: non si diventa membri dell'Unione se se si ricorre alla pena di morte. La Presidenza pertanto si riserva, se necessario, di armonizzare i tempi della discussione della mozione per consentire il rispetto del calendario dei lavori. Così resta stabilito.

Non mi permetto assolutamente di mettere in discussione ciò che delibera la Conferenza dei Capigruppo per quanto attiene ai contenuti, però, signor Presidente, le segnalo che martedì 2 novembre in Italia, pur non essendo una ricorrenza ufficiale,

che, dopo le tante giornate di seduta saltate e perse, non si possa recuperare la ricorrenza dei morti, per chi lo desiderasse (non voglio presumere che ciò valga per tutti), in un altro giorno, lavorativo o non lavorativo, della prossima o di un'altra settimana, francamente mi ha lasciato stupito e un po' allibito. Non credo di essere solitario in questa richiesta, ma sarebbe anche possibile. Ove i colleghi, e soprattutto la Presidenza, lo ritenessero opportuno, nelle forme e nei modi consentiti dal Regolamento del Senato, chiederei la cortesia di rivedere questa decisione,

ho chiesto la presenza del ministro per lo sviluppo economico Romani. Alla luce di quanto dichiarato dall'amministratore delegato della FIAT Marchionne, riteniamo che sia opportuno

In questi giorni il Canton Ticino pubblicizza nell'Italia del Nord - ma le notizie arrivano anche al Sud - la possibilità per le imprese di trasferirsi in Canton Ticino acquistando terreni a tre euro a metro quadro e non pagando le tasse per dieci anni.

i tantissimi dipendenti di piccole e medie imprese che in questi giorni stanno decidendo di chiudere i battenti, qualcuno per trasferirsi e qualcun altro per farla finita dal punto di vista dell'attività buttando sul lastrico l'impresa stessa e soprattutto togliendo occupazione, non solo al Sud, ma in tutto il territorio nazionale.